Avverto che nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna sarà pubblicato l'elenco degli Uffici di Presidenza delle Commissioni permanenti che, in data 21 giugno, hanno proceduto alla propria costituzione.

Ieri il ministro dell'interno Salvini è stato giustamente in Libia per sviluppare accordi volti a frenare l'immigrazione, a fronte dell'emergenza che Italia ed Europa stanno affrontando. Tuttavia, vi è un'altra parte dell'Africa in cui, in questi giorni, sta avvenendo qualcosa di estremamente positivo, purtroppo nella disattenzione del nostro Paese. Mi riferisco al Corno d'Africa, da cui

fatto storico, salutato con estremo favore dalle Nazioni Unite, dall'Unione africana, dall'Unione europea, dagli Stati Uniti e da tanti altri Paesi: Paesi: una delegazione di alto livello del Governo eritreo si sta recando ad Addis Abeba per cogliere le novità che sono venute dall'Etiopia dopo che, in aprile, è stato eletto un vero Governo del cambiamento. *premier* etiope, Abiy Ahmed, ha lanciato un processo di pacificazione e stabilizzazione dell'intera area, anzitutto nei confronti dell'Eritrea, del suo stesso Paese, liberando i detenuti politici, e della vicina Somalia. Questa svolta, di estrema importanza, potrebbe portare finalmente alla pacificazione dell'area,

il nostro Paese. Noi crediamo che questo fatto sia di estrema importanza proprio per i riflessi che può avere sulla stabilizzazione della regione.

Il ruolo dell'Italia nella regione è fondamentale dal punto di vista storico, culturale, economico, politico, strategico, militare e di sicurezza, non solo per l'immigrazione. Noi ci auguriamo che il Governo italiano svolga un ruolo da protagonista non sia assente in un'area di strategico interesse per il nostro Paese. Ci auguriamo altresì che l'Esecutivo spinga l'Unione europea ad assumere, a sua volta, un ruolo da protagonista nella pacificazione e stabilizzazione dell'area, anche attraverso un piano straordinario di sostegno economico e sociale. Insomma,

di rendere un'informativa a quest'Assemblea e, soprattutto, di svolgere un ruolo da protagonista, perché fino a questo momento nessuno se ne è accorto.

all'inizio degli anni 2000, ha fatto un'azione di aiuto e di supporto del nuovo Parlamento somalo che si insediava allora. Eritrea ed Etiopia hanno decine di anni di una guerra guerreggiata che ha portato, per i giovani eritrei, a tre anni di servizio militare obbligatorio; e naturalmente questo ha portato anche a moltiplicare le fughe da quel Paese. Oggi l'iniziativa del Primo Ministro etiopico è di grandissimo rilievo per l'Africa, per il Corno d'Africa e, indirettamente, anche per l'Europa, che da quei Paesi purtroppo vede moltissime persone che arrivano e che

Senatore Casini, vale ovviamente la stessa premura della Presidenza anche per la sua richiesta. Ora, onorevoli colleghi, prima di passare all'ordine del giorno, desidero formulare, a nome di tutti noi, un augurio al senatore Simone Pillon, che è diventato padre di una bambina di nome Elisabetta.

avrebbe potuto, con l'insediamento di un Governo politico, cambiare segno e diventare il veicolo più adeguato per sciogliere nodi che rischiano di rappresentare un ostacolo alla ripresa delle zone dei due crateri sismici. Noi auspichiamo tutto ciò, signor Presidente, ma vorremmo almeno che questo decreto-legge riuscisse a risolvere un problema annoso, che sta avvelenando la vita civile ed economica

Non era mai accaduto che l'epicentro di un terremoto fosse all'interno di una città. L'Abruzzo ha poi un altro triste primato,

Tale specificità dovrebbe essere tenuta presente nel considerare di intervenire su quel che è accaduto e quel che sta accadendo in questa città. Facciamo una piccola cronistoria. In passato in Italia gli interventi a favore delle zone colpite da catastrofi non sono mai stati notificati

ha chiesto agli imprenditori, agli artigiani, ai cittadini che si sono adoperati durante la ricostruzione, di restituire gli sconti avuti, maggiorati dagli interessi. Bisogna poi tener conto che questo è stato fatto solo per L'Aquila. Tutte le mancate notifiche precedenti sono cadute, per così dire, in prescrizione gli interventi successivi a favore delle popolazioni colpite dal sisma nel 2016 e nel 2017 non sono stati considerati aiuti di Stato. Quindi si è venuta a determinare di Stato. Quindi si è venuta a determinare una sorta di finestra di "disopportunità", che riguarda soltanto la città di L'Aquila e il cratere del 2009.

definire scolastica e rigida è dir poco. Qualcuno in quest'Aula mi deve dimostrare che un imprenditore che ha gestito la sua impresa a Monaco oppure a Parigi in questi anni è stato sfavorito per la situazione nella quale si sono venuti a trovare gli imprenditori aquilani, che hanno portato avanti la propria attività in presenza di un vero e proprio disastro.

A meno che noi non aderiamo a una visione quantomeno manichea, che è quella che viene riportata all'interno dell'ordinanza

«un'impresa diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che un aiuto sia stato notificato». Fine della citazione. Qui siamo al paradosso. Colleghi, fondamentalmente l'Europa ci dice non solo coloro i quali hanno fatto impresa a L'Aquila, il centro storico più colpito in questo millennio, devono restituire i soldi, ma anche che quegli imprenditori, che dovrebbero essere reputati degli eroi se si considera la condizione di contesto nella quale hanno operato, avrebbero dovuto

che copriva il periodo compreso tra il 2008 e il 2011. Quel provvedimento, signor Presidente, è nella finanziaria pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 27 novembre 2011.

la schiena dritta, soprattutto quando si ha ragione. Se quest'Assemblea si presenta con un emendamento approvato all'unanimità e contesta

e dimostrerà nei fatti di considerare i nostri cittadini più sfortunati. Essi non sono delle cavie ma dei cittadini di serie A che meritano ancora maggior rispetto.

onorevoli colleghi, ci apprestiamo ad approvare l'ultimo intervento, in ordine di tempo, volto a fronteggiare l'emergenza e indirizzare la delicata fase della ricostruzione

danni materiali stimati dalla Protezione civile sono oltre 23 miliardi e sono andati ad aggiungersi a quelli già ingenti del 2009 e del 2012. È obiettivo primario del Governo, nostro, di tutti, fornire alle popolazioni colpite dal sisma gli strumenti e il sostegno necessari a garantire il ritorno alla normalità, alla vita e al lavoro antecedenti ai tragici eventi. Tanto è stato fatto finora in tal senso e tanto resta ancora da fare. Abbiamo davanti un quadro normativo estremamente complesso a cui vanno aggiunti ben 61 provvedimenti di ordinanza (35 del commissario straordinario e 26 della Protezione civile). Alle popolazioni che con dignità e determinazione hanno affrontato immani sofferenze voglio dire con chiarezza: siamo al vostro fianco, lo saremo più di ieri, con forte impegno e atti concreti. Anche a livello europeo, specie negli ultimi anni, si registrano interventi volti a rafforzare le capacità di risposta e potenziare la prevenzione e la preparazione alle catastrofi. Il Parlamento europeo, nella propria risoluzione sulla situazione Italia dopo i terremoti, ha evidenziato la necessità di attuare sinergie tra tutti i fondi disponibili per sostenere i territori e le zone rurali con attività agricole, invitando gli Stati membri a investire maggiormente nelle attività di ricerca al fine di prevenire i danni e vigilare sul rispetto delle norme di costruzione antisismica. Poc'anzi dicevo che tanto è stato fatto e tanto - mi permetto di dire - poteva essere fatto meglio. Faro del nostro agire deve essere la tutela dei cittadini e dei territori. Dobbiamo prendere atto della necessità di progettare una politica che sia coerente con le specificità del nostro Paese, responsabile non solo amministrativamente, ma anche culturalmente nei confronti dell'intera umanità, di un patrimonio storico, culturale e paesaggistico unico al mondo. Per andare incontro alle esigenze delle popolazioni interessate, la Commissione - che ringrazio - ha, tra le altre cose, ha approvato un emendamento che riapre la finestra temporale per escludere dalla formazione del reddito imponibile i redditi dei fabbricati distrutti: una misura di buon senso, mirata ad alleggerire l'altrimenti insostenibile pressione fiscale. Nel corso dei lavori è stato inoltre approvato un importante ordine del giorno sulla microzonazione sismica, tematica che riveste un ruolo importante e chiave nelle strategie di prevenzione e mitigazione del rischio. da parte del Governo di altri ordini del giorno - ho partecipato ad un paio di sedute della Commissione speciale - riguardanti il potenziamento delle attività e dei percorsi di assistenza psicologica e le agevolazioni fiscali per le imprese che assumono soggetti residenti nei Comuni colpiti. In conclusione, signor Presidente, voglio porre l'accento su alcune sollecitazioni che continuano ad arrivare dalle popolazioni colpite come garantire la massima qualità della ricostruzione, dare continuità al meccanismo di incentivazione per le ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche ed estenderlo anche ad adeguamenti e consolidamenti antisismici. Un'altra richiesta è quella di aggiornare la carta geologica d'Italia e dare il massimo sostegno alle imprese e all'occupazione di tutte le zone colpite. Reputo che, come uomini e donne impegnati nella gestione della cosa pubblica, non possiamo assolutamente permetterci di ignorare questi suggerimenti suggerimenti che arrivano da chi ha visto stravolta la propria esistenza. È nostro dovere ascoltare, nostro compito dare delle risposte efficaci. Io penso, e così pensiamo tutti, di aver fatto, con le con le modifiche che abbiamo proposto al testo del decreto-legge, proprio questo: sostenere la ricostruzione tanto dei luoghi quanto delle aspirazioni delle popolazioni colpite. Sarà un banco di prova, sottosegretario Santangelo, proprio di questa legislatura appena iniziata. Stiamo facendo la nostra parte. L'ottimo lavoro svolto dal relatore Patuanelli, dal collega della Lega Paolo Arrigoni, dal presidente della Commissione Erica Rivolta e soprattutto

di legge n. 435** Il decreto-legge al nostro esame è stato emanato a seguito di ripetute richieste avanzate dalle comunità locali e dalle categorie del settore coinvolte nelle procedure amministrative per la realizzazione degli interventi di ricostruzione post-sisma. Purtroppo, a distanza di due anni dal devastante terremoto che ha colpito il Centro Italia, la ricostruzione non è stata ancora avviata e la popolazione colpita,

procedure lente, vincoli e intoppi burocratici rendono difficoltosa l'approvazione dei piani attuativi. Per avere un'idea degli effettivi ritardi in corso, basti pensare che la rimozione delle macerie non è stata ancora conclusa e che non tutte le "casette" SAE sono state ancora consegnate agli aventi diritto. D'altra parte, l'annuncio dell'arrivo di un decreto-legge sul terremoto 2016-2017 ha creato molte attese da parte di tutti, anche perché i primi testi elaborati dal Commissario per la ricostruzione, con un contenuto composto da 18 articoli, entrava nel merito di una serie di questioni urgenti segnalate dai territori terremotati.

Pertanto, la Commissione speciale si è trovata costretta ad integrare il testo del decreto per rispondere ad una serie di rilevanti richieste di carattere tecnico segnalate dai soggetti auditi, anche se

Proprio per questo, come diceva il collega Castaldi, in Commissione abbiamo scelto insieme di usare un un metodo di lavoro molto serio e approfondito. Abbiamo audito tutti e abbiamo cercato di estrapolare ogni problematica da risolvere.

quindi è da leggere davvero con la massima attenzione e il massimo rispetto per questa terra e, soprattutto, per la popolazione che la abita. *(Applausi dal alcuni emendamenti approvati, promossi dal nostro Gruppo, e prima di tutti un intervento importante sia sulla normativa edilizia, che su quella del codice dei beni culturali e del paesaggio, diretto a permettere l'installazione di manufatti temporanei in aree di proprietà privata nei comuni terremotati, come strutture prefabbricate o amovibili, utilizzati in sostituzione dell'abitazione principale dichiarata inagibile. La norma più volte proposta e sostenuta dalla Lega durante l'esame di precedenti decreti-legge sul terremoto 2016-2017, intende risolvere le situazioni in corso conseguenti allo stato di emergenza provocato dal terremoto del Centro Italia

delle ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e delle misure di sequestro preventivo già emanate per tutti i lavori e le opere che rispettino una serie di condizioni prestabilite. Un'altra questione importante riguarda la possibilità per le diocesi di realizzare interventi fino a 500.000 euro basandosi sulle procedure previste per la ricostruzione privata, che senz'altro permetterà la celere ricostruzione di piccoli lavori nelle chiese terremotate. ricostruzione è la mancata definizione dei condoni passati - e quindi la mancanza di abitabilità e agibilità dell'edificio terremotato per carenza documentale

di avere tutto il nostro aiuto per poter ripartire. Io non penso che i nostri concittadini di queste zone sfortunate non abbiano voglia di ripartire o non abbiano il coraggio. Hanno delle ferite che non saranno mai più rimarginabili, ma bisogna dar loro la possibilità di farlo, dobbiamo necessariamente operare delle semplificazioni,

Io penso che queste persone siano disponibilissime a fare ancora sacrifici, ma con la prospettiva e con con l'obiettivo finale di ricostruire le loro case, di ricominciare le loro attività, di ridare la possibilità ai turisti di godere di queste zone bellissime.

deve emergere questo, poi ci sarà la seconda lettura alla Camera. È stato dimostrato in Commissione speciale e spero venga dimostrato oggi e nei giorni prossimi in quest'Aula, abbiamo il dovere morale, oltre che politico, di dare delle risposte a questa gente. Lo meritano e noi tutti ci dobbiamo impegnare profondamente perché ciò avvenga. È una questione di giustizia.

colleghi, innanzitutto vorrei ringraziare il senatore Patuanelli, relatore del provvedimento, e, allo stesso tempo, mi corre l'obbligo di esprimergli la mia solidarietà, perché immagino l'imbarazzo che abbia provato nel redigere questo documento, perché in esso non vi è nulla: nulla di questo documento inciderà sulla qualità di vita dei nostri concittadini, che da due anni attendono di poter ripartire

la Commissione abbia cercato con grande impegno, ma purtroppo senza successo di trovare una soluzione ai problemi delle piccole difformità. Il relatore ha aggiunto che «Ci sono dei temi che non siamo riusciti a toccare e dei problemi che non siamo riusciti a risolvere», «Dovrà essere fatta una riflessione urbanistica sulla ricostruzione ampia». Poi alza bandiera bianca, quando afferma che le trenta tematiche affrontate non risolvono un solo punto di quelli che ostacolano la partenza della ricostruzione.

sono totalmente contraddittorie e non c'è un riferimento normativo unico. Pertanto, non presenta la dichiarazione e, pertanto, non si ottengono i contributi e, pertanto, non riparte la ricostruzione.

Temo che ci stiamo dimenticando di chi stiamo parlando. Stiamo parlando di persone che hanno perso una casa, hanno perso una piazza, una chiesa, un lavoro, hanno perso la propria dignità e noi oggi, a distanza di due anni, stiamo dicendo loro di aspettare, perché ancora non siamo capaci di dire loro come si fanno le cose. Questo è intollerabile! E sapete qual è la cosa più grave? Che i soldi ci sono: ci sono i finanziamenti pubblici; ci sono i fondi europei. Il presidente del Parlamento europeo Tajani - che ringraziamo per i suoi buoni uffici - ha annunciato che ci sono un sacco di soldi, dalla vituperata Europa, eppure i progetti non partono. Presidente, a volo pindarico perché il tempo è assai ristretto, vorremmo evidenziare alcune contraddizioni che potevano essere cancellate subito. Si immagini che a distanza di due anni non si è cancellata quella sperequazione di trattamento tra coloro che abitano nei centri e nelle zone rosse rispetto a chi abita fuori dal centro del borgo. Ormai nessun borgo medievale e nessuna città colpita dal sisma abitanti nel centro, per cui si danno i vantaggi a pochissime persone, perché ormai tutti i borghi medievali sono disabilitati. La gente vive fuori e tutti coloro che hanno costruito fuori per motivi di manutenzione, di qualità di vita o di agevolazioni non possono fruire di alcuna agevolazioni, se non della proroga di alcune facilitazioni in termini fiscali. Noi chiediamo, in sintesi, che si elimini la proroga della scadenza della sospensione dei mutui solo nelle zone rosse perché, ad esempio, Ascoli Piceno ha 800 persone e famiglie evacuate, ma non rientra nelle zone rosse. Si rende conto di cosa stiamo parlando? Non ci voleva molto. L'esenzione del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per le strutture di cantiere è riservata solo alle imprese che operano la ricostruzione nei centri storici. Questa roba potevamo eliminarla. La maggioranza lo poteva fare. Capisco che è difficile in un tempo così ristretto. Non si chiede il cambiamento radicale, ma almeno il cambio del passo e, in fondo, bisogna anche inserire un altro aspetto: è assolutamente necessario definire il limite tra difformità e abuso, per distinguere eventuali nuovi volumi per fini speculativi da quelli volti a rendere fruibili i volumi preesistenti. Vado a concludere, signor Presidente. Penso che ciascuno di noi voglia fare il proprio lavoro dando valore alla politica, se la politica è ancora capace di assumersi delle responsabilità. Qui, oggi, non abbiamo assunto alcuna responsabilità, abbiamo fatto gli amministratori, anzi gli amministrativi, che forse

Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, rappresentanti del Governo, oggi il Senato si appresta a convertire un decreto-legge che cerca di dare risposta ai problemi drammatici delle centinaia di migliaia di terremotati che in quattro Regioni d'Italia hanno perso case, aziende, interi paesi e purtroppo anche i loro familiari. Ebbene, alle vittime innocenti che da Amatrice a Rigopiano hanno perso le loro vite va innanzitutto il nostro pensiero; vittime di una calamità imprevedibile, certo, ma anche dell'inettitudine di chi, alla testa di amministrazioni locali e regionali, avrebbe dovuto mettere in campo tutte le misure necessarie di prevenzione dei rischi. Queste perdite e questi lutti chiamano il Parlamento a un impegno rinnovato e solenne per convertire questo decreto-legge, ma soprattutto per aprire una pagina nuova sul fronte delle catastrofi naturali, e del terremoto in particolare, iniziando a creare le premesse per indirizzi di effettivo cambiamento che non ci impegnino solo a fronteggiare in emergenza i disastri, ma anche e soprattutto a prevenire e ad eliminare i rischi. Il decreto-legge che stiamo esaminando, proposto dal Governo Gentiloni Silveri, era costituito, come è noto, di soli due articoli e ci chiedeva, in pratica, di disciplinare proroghe e sospensioni di natura tributaria e contributiva, compresa la sospensione del pagamento del canone televisivo. Solo questo, insomma, come se per tutto il resto - e il resto sono le condizioni drammatiche in cui vivono le 50.157 persone assistite negli alberghi e in altri alloggi di fortuna non ci fosse l'urgenza di mettere in campo misure di carattere straordinario davvero in grado di avviare una ricostruzione tempestiva ed efficace dei territori colpiti. Con una risposta di straordinario impegno e generosità, la nuova maggioranza di Governo e le altre forze politiche, attraverso la Commissione speciale, hanno fortunatamente allargato lo spettro dei problemi affrontati nel decreto-legge mettendo mano a tantissime delle urgenze dettate dalla situazione disastrosa delle zone calamitate. E così, attraverso i 42 emendamenti approvati che hanno toccato ben 30 - ripeto: 30 - nuove e diverse tematiche, sono state varate misure che, tra le altre cose, prorogano la struttura commissariale e lo stato di emergenza, il pagamento di tasse e tributi; prorogano mutui e indennità a favore dei sindaci, scadenze IRPEF e IRES; prorogano la cassa integrazione; accelerano insomma davvero la ricostruzione. Ricordo anche l'avvio di soluzione che è stato dato alla questione degli sgravi concessi alle aziende colpite dal terremoto di L'Aquila del 2009, dalla Unione europea considerati aiuti di Stato a causa delle

e che occorre focalizzare l'attenzione sull'urgenza della prevenzione. Qualche dato: nel 2016 la rete sismica nazionale ha registrato oltre 53.000 terremoti contro una media annua di circa 20.000; dal 2000 oggi l'INGV ha registrato 39 terremoti di magnitudo superiore a 5 gradi, di cui 10 tra il 2016 e il 2017. E il futuro, purtroppo, non promette niente di buono. Ebbene, cosa stiamo facendo noi di concreto per la prevenzione? Per esempio sappiamo, dato che le statistiche sono impietose, che la gran parte degli edifici scolastici italiani è a rischio

Tutto questo - lo ripeto - in Abruzzo, Regione dei terremoti per eccellenza; lo stesso Abruzzo dove l'esposizione a rischio è massima e indiscriminata, come è successo nel caso dell'albergo di Rigopiano, dove, in occasione dei terremoti di gennaio del 2017 sono morte inutilmente le persone che sapete. Sarebbe bastato che la Regione avesse messo in campo la necessaria carta delle valanghe per evitare la catastrofe, impedendo l'apertura di quella struttura Per queste inadempienze sono oggi indagati per omicidio, lesione e disastro colposo i tre Presidenti di Regione che si sono susseguiti nell'ultimo decennio: Ottaviano Del Turco, Gianni Chiodi e Luciano D'Alfonso, senatore governatore presente in quest'Aula, sebbene in una situazione di acclarata incompatibilità. Ebbene - dicevo - cosa facciamo noi davanti a questa situazione? Da qui ai prossimi venti anni metteremo in campo circa 40 miliardi di investimenti, sono stati stanziati circa 40 miliardi. Dobbiamo capire quello che è successo negli ultimi anni, come sono state impiegate queste risorse e soprattutto prevenire, prevenire e prevenire. È ora che il Parlamento prenda di petto la questione e lo faccia attraverso l'istituzione ad una Commissione d'inchiesta per chiarire anzitutto la situazione di rischio reale nel Paese e avviare un'indagine sull'effettivo impiego di quelle risorse. Soprattutto, però, il tema vero - lo ripeto in quest'Aula e lo griderei ancora più forte - è l'impegno improcrastinabile per la prevenzione e la mitigazione del rischio, senza dimenticare a questo punto un'adeguata messa a fuoco per una politica degli incentivi per interventi di adeguamento e consolidamento antisismico degli edifici pubblici e privati su tutto il territorio nazionale.

Signor Presidente, il presente disegno di legge di conversione prevede - come è noto non solo agli addetti ai lavori, ma in particolare ai diretti interessati, ovvero ai tanti contribuenti delle Regioni coinvolte dagli eventi sismici dell'agosto 2016 - misure per la sospensione dei termini tributari e contributivi. Il provvedimento d'urgenza, in prima lettura al Senato e assegnato alla Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo, come è stato ricordato da chi mi ha preceduto, nasce dall'esigenza di venire incontro alle popolazioni e alle imprese del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) che, successivamente alla giornata del 24 agosto 2016, hanno visto cadere le più ovvie certezze della propria vita quotidiana. Su questa terribile vicenda, con le drammatiche conseguenze che ne sono derivate, ricordo come Fratelli d'Italia sia stata la prima forza politica della coalizione di centrodestra ad aver posto come questione prioritaria quella riguardante il sostegno e l'assistenza alle popolazioni terremotate. Le misure contenute nel provvedimento risultano tuttavia ancora insufficienti ad invertire l'attuale situazione in cui si trova la popolazione coinvolta dal sisma del 2016. al mancato finanziamento dei contratti a termine, in scadenza dicembre, che riguardano figure tecniche e amministrative importanti e necessarie per continuare le opere di ricostruzione, all'assenza di risorse da destinare alle circa 700 unità di personale che stanno già lavorando nei 130 Comuni del cratere o quelli in deroga per le assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale, in cui i costi saranno a carico dei già precari bilanci comunali. Sono solo alcune misure che, a mio avviso, avrebbero dovuto trovare spazio all'interno del testo e che avrebbero consentito una più celere attività del ripristino delle condizioni di normalità. La necessità di intervenire, pertanto, anche in seconda lettura alla Camera, per non correre il rischio di bloccare le procedure di ricostruzione avviate, anche alla luce della modifica approvata dalla Commissione speciale che assegna ai Comuni il compito di svolgere le attività istruttorie per il rilascio del parere di conformità ambientale e urbanistica rispetto alle opere di ricostruzione, credo possa essere un percorso legislativo da condividere, considerando che il decreto-legge scade il 29 luglio. Venendo agli interventi positivi, non posso non segnalare con favore la previsione di una proroga dei mutui dei Comuni coinvolti dal sisma, anche se andrebbe specificato che detta proroga si applica a tutti i mutui contratti dai Comuni del cratere indipendentemente dal soggetto con cui questo è stato assunto: per quelli contratti con Cassa depositi e prestiti, come attualmente previsto. Pertanto, il decreto-legge nel suo complesso affronta aspetti indubbiamente emergenziali, indifferibili, come testimonia la sua natura di emergenza. Ma al tempo stesso emerge la necessità di garantire ai sindaci dei Comuni coinvolti più potere di intervento diretto e più e più risorse, affinché le tristi esperienze del recente passato, caratterizzate da gestioni dei precedenti Governi superficiali e pasticciate, possano finalmente essere solo un ricordo lontano. In sostanza, nel complesso si evince un tessuto legislativo del provvedimento che è composto da due soli articoli, cui si è aggiunto successivamente, nel corso della fase emendativa della Commissione speciale, la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2018, con l'auspicio che nei prossimi provvedimenti all'esame del Parlamento si preveda nella legge di bilancio di prorogare ulteriormente la scadenza. Questo è un auspicio e speriamo che possa accadere. Ciononostante, il mio avviso è che uno sforzo in più da parte del Governo per venire incontro alle popolazioni e alle imprese coinvolte del sisma si sarebbe potuto fare. Penso agli sgravi sulle assunzioni, al potenziamento degli uffici speciali, alla ricostruzione e ad altre agevolazioni. Misure che sono state trasformate in ordini del giorno non vincolanti oppure rinviate, con genetiche premesse di interventi, a non prima di settembre. A quasi due anni dal primo sisma che ha devastato il Centro Italia il quadro normativo in materia di ricostruzione risulta molto articolato e complesso. Pensiamo soltanto che sono state fatte 56 ordinanze commissariali e un numero altrettante grande di ordinanze del capo dipartimento della Protezione civile che stenta a produrre risultati concreti in termini di ricostruzione. difficoltà di avvio della ricostruzione, su cui ha pesato e continua a pesare l'eccessiva complessità delle procedure, occorrono semplificazioni in grado di accelerare realmente il processo di ricostruzione. Termino, signor dicendo che noi, come Fratelli d'Italia, incalzeremo il Governo affinché dimostri di fare meglio del precedente, perché si può fare molto meglio, come fece un altro Governo che non lontano da qui, a L'Aquila, dimostrò che le case temporanee erano temporanee e non soltanto definitive.

*(PD)*. Signor Presidente, cari colleghi, spero che ci sia la dovuta attenzione. Un ringraziamento va anche al rappresentante del Governo. Io non credo che questa sia solo una discussione di facciata; voglio ritenere che questa discussione sia un investimento di intelligenza da parte di tutti per arricchire e strutturare la la forza del decreto-legge che ci apprestiamo a convertire in legge, soprattutto per onorare anche il lavoro che abbiamo fatto in Commissione speciale. Questo prodotto normativo si è posto sostanzialmente tre problemi. Il primo problema riguarda lo spostamento delle scadenze in avanti, a cominciare dall'importante scadenza riguardante la gestione delle emergenze e vorrei invitare i colleghi che hanno parlato e quelli che parleranno a cogliere l'effettività di due fasi che entrano in campo quando c'è una emergenza da disastro. C'è il primo intervento, che ha carattere emergenziale, e poi si dà luogo alla ricostruzione. Noi stiamo cercando di dare ulteriore copertura normativa alle esigenze della ricostruzione, per la quale esiste copertura finanziaria all'altezza e per la quale sappiamo che vi sono un canale di ricostruzione delle opere pubbliche e di pubblica utilità e un canale riguardante la ricostruzione privata.

una vicenda problematica ancora non affrontata in modo adeguato, vale a dire la piccola e lieve difformità urbanistica che, se non affrontata in termini esaustivi, non consente la procedimentalizzazione dei contributi riferiti alla ricostruzione privata. Dunque, un lavoro in Assemblea di questo tipo e il lavoro fatto con onestà intellettuale in Commissione speciale non devono dar luogo ad un'ipocrisia cartacea: devono dare luogo ad un'adeguatezza normativa che consenta poi adeguatezza amministrativa da parte degli enti locali. Noi sappiamo che le piccole difformità non stanno rallentando, stanno bloccando la ricostruzione privata. Non può essere il ritenere ideologicamente sbagliato entrare nel merito ciò che ci impedisce di entrare nel merito di una soluzione a portata di mano: fare le audizioni, incontrarsi, scrivere articoli e discutere anche qui dentro e poi non dare luogo ad un prodotto all'altezza dell'esigenza normativa significa ipocrisia e immoralità. C'è poi la terza questione, riguardante la ripresa di vitalità economica delle imprese. Noi non dobbiamo ricostruire città di mura che assomigliano a cimiteri; noi dobbiamo ricostruire città

che, da una parte, hanno ricevuto ausilio e aiuto e che, dall'altra, adesso subiscono e vedono un atteggiamento sanzionatorio, afflittivo, che chiede un recupero e non si tratta di un recupero che deve partire domani o dopodomani, ma che è già procedura dell'Agenzia delle entrate con un commissario *ad acta*.

cogliamo questa occasione. Qui si sta svolgendo e ha luogo un confronto dialogico che deve nutrire il merito del lavoro. Mi auguro che questo intervento, come quelli degli altri, possa aiutare il prodotto finale che serve a quei territori per ricominciare a vivere.

*(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, siamo ad un nuovo appuntamento con un decreto-legge terremoto, un tema che

importante, in uno spirito di collaborazione che, in linea di principio, porta rispetto a tutte quelle persone che stanno aspettando dunque è un fatto nuovo, un fatto importante, che riguarda un decreto-legge che è nato a cavallo non tra due legislature, ma tra due Governi, con sostanziali cambiamenti, perché il Governo che

dalle forze di minoranza, ma sono stati approvati all'unanimità. Ribadisco questo concetto, per testimoniare il grande spirito di collaborazione, non soltanto tra le forze che in questo momento sono parte della

Abbiamo affrontato vari temi e chiaramente il tema del terremoto è estremamente complesso e noi che veniamo da quelle zone sappiamo quanto sia complesso sul terreno, ma anche a livello normativo.

l'emergenza terremoto è stata affrontata, purtroppo, in maniera emergenziale, il che significa che non ci siamo fatti trovare pronti per questo evento estremamente drammatico, che pure è andato al di là delle

ad esempio, di adeguamento sismico delle scuole o di altri uffici pubblici, ciò ci fa capire che, probabilmente, la strada da percorrere è ancora molta e va percorsa nel

colleghi senatori, qui ho sentito parlare di persone che hanno perso casa, di persone che hanno perso il lavoro, di partite IVA senza futuro. Ho sentito parlare di tante problematiche e rientro in ciascuna di esse. Da sindaco di uno dei Comuni terremotati e da cittadino di uno dei Comuni distrutti credo che nessuno più di me possa volere tutto e subito, quando si parla di terremoto. Tutto e subito, però, e non è possibile lo sappiamo bene. Il decreto-legge in esame, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, in realtà conteneva solo poche proroghe fiscali.

non è la forma corretta, perché in realtà le scosse continuano ancora. Lo sciame sismico che ancora colpisce l'Italia centrale è un fenomeno che non ha precedenti nella storia recente dell'Italia e ha pochi precedenti nella storia millenaria della nostra nazione.

frane hanno interrotto strade anche di interesse nazionale, fiumi hanno visto aumentare la loro portata fino al triplo della media del periodo, perché la rottura delle sacche sotterranee ha fatto sì che il rilascio contestuale di quella gran massa d'acqua abbia gonfiato tutti i fiumi della zona. Un fiume scomparso da decenni ha ricominciato a scorrere. In uno dei luoghi più suggestivi d'Italia, Castelluccio di Norcia, si sono formate voragini sul terreno e nel fermano si sono creati vulcanelli di fango. I numeri possono forse dare la misura di quello che è successo, ma nulla può dare la dimensione dell'angoscia provata da chi ha perso tutto, la propria casa e il proprio futuro. Ecco perché ritengo necessaria questa premessa, perché oltre alle conseguenze che abbiamo ben chiare, viste in tantissimi servizi televisivi, sull'ambiente naturale e sui Comuni, ci sono state conseguenze sulle persone: conseguenze fisiche, con centinaia di feriti e, purtroppo, numerosi morti, ma anche conseguenze psicologiche, non tutte a causa diretta del terremoto. Non ci dobbiamo nascondere che il dramma che ha colpito quelle popolazioni e, soprattutto, la perdita di speranza

La domanda che ora dovremmo porre e porci tutti noi è: perché le persone hanno perso la speranza? Se facessimo questa semplice domanda a qualunque residente di quei territori la risposta sarebbe sempre la stessa: ci avevano promesso che non saremmo stati abbandonati e invece lo Stato ci ha lasciato soli. Questa è sicuramente la risposta più comune che riceveremmo, ma non è una risposta vera, perché i Vigili del fuoco non hanno abbandonato nessuno, perché l'Esercito non ha abbandonato nessuno.

la stragrande maggioranza delle persone sente di essere stata abbandonata è perché è mancata la politica. Siamo mancati noi. *(Applausi È mancato chi si prendesse la responsabilità di decidere come poter ricostruire secondo l'esigenza più importante di quelle persone: persone: tornare a casa propria in tempi rapidi e ricostruire il proprio futuro. È questo quello che oggi vorrei evidenziare e che serve a mio avviso di più in assoluto in questa ricostruzione: serve che le persone vengano rimesse al centro dell'attenzione. Così non è. Da subito si è dichiarato che sarebbe stata prioritaria la legalità, da subito si è dichiarato che sarebbero stati prioritari i tempi, da subito si è dichiarato che sarebbe stato prioritario individuare un metodo di ricostruzione. Ma mai si è detto che sarebbe stata prioritaria la ricostruzione, che era l'elemento necessario a quelle persone per recuperare la speranza. La rapidità, elemento fondamentale, non l'abbiamo mai riscontrata, nemmeno nella gestione dell'emergenza: un assurdo. Per definizione l'emergenza dovrebbe risolversi nell'imminenza del fatto; invece sono passati quasi due anni dal terremoto e molte diverse centinaia, ancora non sono state consegnate, perché erano necessari nove passaggi per la loro realizzazione. Molti hanno evidenziato il costo notevole, enorme, di quelle realizzazioni, io voglio evidenziare invece il fatto che che sono state realizzate in un tempo del tutto inaccettabile per la gestione di un'emergenza. Però queste non sono le uniche difficoltà riscontrate, perché anche nella gestione della ricostruzione troviamo un'analoga situazione. Qualche settimana fa è stata gettata la prima pietra per la ricostruzione della scuola di San Ginesio, ricostruita direttamente dalla struttura commissariale. Dopo pochi giorni anche quella ricostruzione si è bloccata, perché nemmeno lo stesso commissario speciale per la ricostruzione, con questa situazione, riesce a ricostruire. Non riescono a farlo i Comuni, che si trovano purtroppo impelagati in una burocrazia quasi impossibile da superare, non riescono a farlo i privati, che vorrebbero trovare soddisfazione da soli alle proprie esigenze, non riescono a farlo nemmeno gli altri soggetti, che hanno tentato in qualche modo di accelerare la ricostruzione, e non ce la fa nemmeno lo stesso commissario: una scuola ricostruita dal commissario è stata immediatamente bloccata. Arriviamo quindi al fallimento totale di questa impostazione. Lo strumento principe della ricostruzione dei Comuni distrutti, i piani attuativi predisposti dopo perimetrazioni delle zone maggiormente danneggiate o con un particolare pregio architettonico delle stesse, dopo mesi che dovevano partire sono tutti fermi al palo. Io, da sindaco, sabato prossimo proporrò al mio Consiglio comunale l'uscita dalle perimetrazioni. Quello che doveva essere lo strumento di supporto più importante per la ricostruzione non solo non è stato l'opportunità che doveva essere, ma è diventato addirittura un ostacolo. Se tutto questo è stato fronteggiato dal pubblico, allora qual è la situazione per i privati? Beh, è facilmente intuibile. L'unico modo per superare tutto ciò è che, al bivio in cui ci troviamo ora, la nostra scelta non sia quella di continuare secondo le modalità già definite che hanno portato a quel quadro di sconforto e di disperazione che abbiamo riscontrato fino ad ora; occorre che ci si prenda la responsabilità di fare delle scelte. E la prima scelta è quella di superare il problema delle difformità. Io però non voglio ricorrere ad artifizi verbali, perché in Italia, se uno chiude una scala o realizza una villa in riva al mare, sempre di abuso edilizio si tratta; serve quindi il coraggio di sfatare i tabù: se dobbiamo se dobbiamo parlare di sanatorie riguardo a queste difformità, dobbiamo prenderci la responsabilità di farlo, perché la ricostruzione dei Comuni distrutti avverrà per aggregati ed è sufficiente una piccola difformità in un aggregato per bloccare tutta la ricostruzione. Colleghi senatori, dobbiamo sbloccare le pratiche e, per sbloccare le pratiche, ci dobbiamo prendere la responsabilità di fare la cosa giusta. La cosa giusta è superare certe ipocrisie, sfatare certi tabù

Il valore economico di quegli edifici è tale per cui non si arriva quasi mai a superare la metà del loro costo materiale di realizzazione. Non stiamo parlando di speculazioni, non stiamo parlando di un vantaggio patrimoniale, non stiamo parlando di un vantaggio economico avuto da chi ha realizzato quelle difformità; parliamo di necessità soddisfatte negli anni, in maniera evidentemente irregolare, ma a cui bisogna porre rimedio, altrimenti quelli che sono certificati come i borghi più belli d'Italia, quelle che sono bandiere arancioni del Touring Club, Comuni che rientrano in Parchi nazionali non saranno ricostruiti. È questa, infatti, la realtà; non siamo in presenza di un'anarchia totale o di una degenerazione dell'ambiente causata dall'uomo, ma siamo in luoghi riconosciuti di pregio in tutta Italia e noi abbiamo il dovere,

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, dice la saggezza popolare che è nel momento del bisogno che si riconoscono gli amici e credo che questo sia vero, come credo sia vero che è nel momento eccezionale che si riconosce la tempra di cui è fatto uno Stato e la qualità di una classe dirigente, che ricopre, più o meno fortunosamente, le funzioni di Governo. Governo. Non c'è nulla di più straordinario e devastante di un terremoto. Sono passati quasi due anni dalla prima scossa che ha spezzato in due l'Italia e sono passati invano: le macerie sono in buona parte ancora riverse al suolo, come erano riverse al suolo un'ora dopo il sisma; le mitiche casette, per altro inadeguate ai climi rigidi dell'Appennino, sono in buona parte ancora da consegnare; i centri storici cittadini sono ancora chiusi; le pratiche sono in buona parte ferme o procedono a rilento. Allora, forse è bene ricordare tutti che sotto quelle macerie sono morti 300 italiani. Sarebbe opportuno, se ci fosse il tempo, qui, oggi, ricordare i nomi, i cognomi e le storie di ciascuno di loro. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. E le storie di ciascuna delle famiglie, delle decine di migliaia di famiglie di nostri connazionali che in questo preciso momento e da due anni a questa parte vivono nella condizione di sfollati, lontani dalle loro radici, dalle loro case, dai loro affetti, dai loro lavori e, per i più piccoli, lontani dalle scuole. Tutto questo è inammissibile, è una tragedia nazionale, che la Nazione ha compreso perfettamente da subito. C'è stata una meravigliosa gara di solidarietà per portare sostegno e aiuto alle popolazioni colpite. alle popolazioni colpite. Tutte le popolazioni colpite hanno dato a noi una dimostrazione straordinaria di dignità e di stoicismo: i cittadini del Lazio, quelli dell'Abruzzo, tutti i cittadini e quelli delle Marche in modo particolare (mi si consenta dirlo, perché le Marche sono state la Regione più colpita, la più dimenticata e, ad oggi, la peggio governata da questo punto di vista). La Nazione ha fatto il suo dovere; lo Stato, invece, no. Lo Stato era ed è latitante. *(Applausi dal al contratto sociale, quel patto implicito che lega i cittadini alle istituzioni, in ragione del quale i cittadini rinunciano a una parte della propria libertà e, in cambio, ottengono sicurezza e protezione; quella sicurezza e quella protezione che non sono stati, ad oggi, ancora garantiti ai nostri concittadini colpiti dal terremoto. Questo è inaccettabile. Uno Stato degno di questo nome non abbandona i propri cittadini; uno Stato come l'Italia non può assistere passivamente all'inesorabile - inesorabile, ripeto - spopolamento di piccoli Comuni, perché i piccoli Comuni sono la nostra identità e la spina dorsale di questo Paese. Sarebbe inutile ora mettersi a rivangare gli errori del passato, l'ottuso e scellerato smantellamento della Protezione civile, costituita dal Governo Berlusconi, non per scelta razionale, ma per furore ideologico. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Le promesse da marinaio fatte da presidenti del Consiglio inclini al narcisismo (lo dico per inciso: mi dispiace constatare l'assenza del senatore Matteo Renzi oggi in quest'Aula). Pensiamo al futuro, non pensiamo al passato, cerchiamo di ricucire questo strappo tra la Nazione e lo Stato, perché questo strappo delegittima le istituzioni, noi stessi. Lo Stato non è più credibile se non sarà in grado di portare sollievo velocemente alle popolazioni colpite. Forza Italia ha presentato più di 100 emendamenti in Commissione speciale, tutti studiati con i nostri amministratori locali, tutti calibrati sulle esigenze reali dei cittadini. Alcuni sono stati approvati - e questo è un bene - altri sono stati respinti, altri ancora trasformati - e questa sembra un po' una beffa - in ordini del giorno. Il sottosegretario Laura Castelli si è assunta la responsabilità di non accettare alcuni emendamenti fondamentali; ne dico solo uno, ma sarebbero tanti, ovvero quello che prevede di stabilizzare e prorogare i contratti per circa 700 funzionari chiamati a sostenere le amministrazioni dei piccoli Comuni per mandare avanti le pratiche. Colleghi, se quei contratti non vengono ripristinati, è la paralisi; il resto sono chiacchiere, velleità. quindi, assolutamente provvedere, e - parlo ai rappresentanti del Governo - se il cambiamento che vi siete intestati e di cui avete fatto una bandiera non è solo propaganda, se non è solo retorica, ma una reale spinta per segnare una cesura -auspicabile - tra il passato e il presente, in vista di un futuro migliore per i nostri concittadini, ebbene, questo cambiamento deve essere operativo subito. Occorre siglare un patto tra le istituzioni, il Parlamento e il Governo, indipendentemente dalle appartenenze politiche e dai partiti di appartenenza, affinché questo *vulnus* venga sanato, affinché questa grave ferita nella carne viva della Nazione venga ricucita. Occorre volontà politica, occorrono risorse. Forza Italia la volontà politica ce la mette tutta; le risorse, però, dovete metterle voi del Governo del cambiamento.

che, firmando questo decreto-legge, hanno dimostrato per l'ennesima volta grande attenzione e sensibilità nei confronti delle problematiche del terremoto. E, ancora, ringrazio l'onorevole Paola De Micheli, commissario per la ricostruzione, per il grande lavoro fatto anche in questa fase di confronto e condivisione con tutti i Gruppi parlamentari, oltre che i Presidenti delle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Vorrei ringraziare infine i colleghi senatori del Gruppo per la competenza e l'attenzione con cui hanno seguito i lavori in Commissione speciale e poi in Il provvedimento che stiamo discutendo contiene un pacchetto di norme urgenti introdotte per evitare che venissero meno una serie di agevolazioni previste per le aree terremotate del Centro-Italia, e risulta arricchito dal lavoro della Commissione speciale. È un decreto-legge di manutenzione dei provvedimenti precedenti, che deve accompagnare e migliorare le azioni intraprese. Risulta fondamentale la decisione relativa alla proroga dello stato di emergenza per le aree terremotate fino al 31 dicembre 2018. Vanno evidenziati i provvedimenti volti al sostegno al reddito, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti dei versamenti tributari fino al 16 gennaio 2019, così come la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali fino al 31 gennaio 2019.

per gli interventi di immediata esecuzione, la revisione della soglia di obbligatorietà delle SOA per le imprese, la semplificazione delle procedure di compatibilità urbanistica, così come la proposta di salvaguardia rivolta a coloro che hanno adottato soluzioni autonome con manufatti e strutture nei terreni in prossimità dell'immobile distrutto o danneggiato (la famosa «questione di nonna Peppina»). Ancora, le importanti norme a favore dei Comuni, tra cui l'inserimento degli stessi come soggetti attuatori degli interventi pubblici, la proroga delle scadenze dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e la semplificazione per l'individuazione del responsabile unico del procedimento (questione complessa per le amministrazioni comunali). Da sottolineare è, poi, l'attenzione riposta in materia ai provvedimenti di sostegno al reddito dei lavoratori delle aziende in crisi con più di 400 unità lavorative, ubicate nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e comprese nelle aree riconosciute come di crisi industriale complessa. Questo quadro di riferimento ci consente una riflessione complessiva sullo stato dell'arte. Il bilancio degli eventi sismici del 2016-2017 è stato pesantissimo in termini di vite umane e di economia del territorio, con una stima approssimativa dei danni e dei costi causati dal terremoto che ammonta a oltre 23,5 miliardi di euro. A partire dall'agosto 2016 sono stati stanziati per il sisma 13,16 miliardi di euro di cui 6 miliardi dedicati alla ricostruzione, cifra mai stanziata per una ricostruzione. In questo decennio il terremoto economico provocato dalla crisi globale ed europea ha messo a dura prova l'Italia. La ripresa è cominciata grazie alla solidità del tessuto familiare e alla capacità di resistere e rilanciarsi di molte imprese. Occorre lungimiranza nelle scelte, consolidare le molte riforme strutturali già fatte, continuare sulla strada tracciata per aiutare il sistema produttivo ad affrontare con successo le grandi sfide dell'economia mondiale contemporanea. Il terremoto fisico ha colpito duramente il nostro Paese, soprattutto i nostri territori dell'Appennino centrale, come purtroppo altre parti dell'Italia in passato. Pertanto, anche in questo campo sono necessari previdenza e lungimiranza nelle scelte. Con il provvedimento che oggi discutiamo vogliamo dare solidità a tali scelte perché siamo convinti che esse vadano consolidate e, laddove sia utile, perfezionate. I territori colpiti dal terremoto sono, per giudizio comune, tra quelli più dotati di civismo di capitale sociale. Secondo molti esperti, ciò ha contribuito alla loro prosperità grazie allo sviluppo dei sistemi locali di piccole imprese e adesso deve e può aiutare la loro evoluzione intelligente a fronte dei mutamenti in atto. conclusione, la ricostruzione è dolorosa, è una urgente necessità di oggi ed è anche una sfida aperta per il futuro più lontano. Il terremoto è un dramma, ma non è una condanna al declino e provare a lavorare insieme su questo obiettivo, senza propaganda e polemiche strumentali, sarebbe il modo migliore per dare al nostro Paese la fiducia e la forza che merita.

il provvedimento discusso oggi, rivolto alle famiglie e alle imprese dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, è finalizzato ad una proroga degli adempimenti fiscali per consentire il varo di misure strutturali più complesse volte alla ricostruzione dei centri danneggiati e alla ripresa di quelle attività economiche e sociali che danno origine al dovere di contribuire fiscalmente all'economia generale del Paese. È palese che alla sospensione agevolata dei termini il Governo precedente non ha dato seguito con le necessarie azioni in grado di rimettere letteralmente in piedi i luoghi e le persone coinvolti negli eventi sismici. Spetta a noi, allora - partendo dall'ipotesi che il terremoto non sia avvenuto due anni fa ma ieri, in quanto nulla di concreto ancora è stato fatto provvedere ai bisogni di queste popolazioni, ripartendo da azioni propedeutiche non solo alla ricostruzione ma addirittura agli interventi di messa in sicurezza. Permettetemi di aprire una breve parentesi sulle questioni che in questi giorni stanno infiammando la discussione tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea, ma soprattutto tra le stesse forze politiche del nostro Paese, di maggioranza e opposizione. Se è vero, com'è vero, che il popolo italiano vanta, e ne è fiero, proprio in base alla nostra Carta costituzionale, una tradizione di solidarietà verso qualsiasi individuo e situazione di difficoltà, ancora maggiore attenzione, solidarietà, preoccupazione e impegno andavano e vanno rivolti verso i nostri connazionali vittime di eventi sismici non solo di Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche che da anni ormai vivono in condizioni di precarietà, subendo - oserei dire - una condizione di subalternità alle esigenze del sistema di *business* sull'immigrazione cosiddetta economica. Queste popolazioni, dal momento cronologico dell'evento ad ora, continuano a vivere e a rimanere in uno stato di immediato *post* terremoto. Oggi, 26 giugno 2018, oltre alla necessità di prorogare ed integrare i termini relativi agli adempimenti di natura fiscale e tributaria, grazie agli emendamenti inseriti, sono stati previsti la proroga dello stato di emergenza con quantificazione dei relativi oneri finanziari, la creazione di aree attrezzate per finalità turistiche e le concessioni di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata con interventi di adeguamento alla normativa antincendio e igienico-sanitaria nonché per l'eliminazione delle barriere architettoniche. procedure concorrenziali di affidamento per una ricostruzione più rapida dell'enorme patrimonio culturale ecclesiastico ancora inagibile, indennità di occupazione di suolo pubblico, semplificazione amministrativa. Come è emerso nel corso delle varie audizioni in Commissione speciale, la contrazione delle attività economiche ha comportato, non soltanto nelle zone del cosiddetto cratere, una significativa riduzione del prodotto interno lordo, indebolendo il già fragile sistema economico locale, con un evidente peggioramento delle condizioni di qualità della vita. Esattamente una settimana fa, proprio in quest'Aula, abbiamo dato il via libera al DEF 2018 e nel quadro programmatico si dovrà necessariamente intervenire con scelte politiche più forti, incisive, coerenti e concrete, che consentano di tenere attivi i processi produttivi esistenti in queste aree per rilanciarli in termini di competitività e sviluppo. Di fronte alle emergenze, lo Stato deve intervenire in tutte le sue articolazioni, garantendo efficienza ed efficacia di soluzioni e pur apprezzando il valore insostituibile dei tanti volontari, ritengo sia necessario un potenziamento numerico e strumentale delle nostre Forze dell'ordine e soprattutto del Corpo dei vigili del fuoco, interessati da più anni, ormai, da notevoli carenze di organico e da forti penalizzazioni economiche che un Paese civile socialmente evoluto non può e non deve assolutamente consentire. Assume anche una particolare evidenza la questione degli enti locali, dopo il disastro causato da chi ha pensato di riformare le amministrazioni locali, snaturandone il ruolo, tagliando i fondi e lasciandone però immutate le competenze. Mi riferisco, in particolare, alla riforma Delrio, ovvero alla scellerata imposizione di una riforma monca che ha reso le Province, enti essenziali a ridurre la distanza tra lo Stato e i territori, impossibilitate ad adempiere alle loro funzioni, ma mantenendone una struttura mastodontica, senza contare la spoliazione del diritto di scelta politica amministrativa, che noi cittadini esprimevamo attraverso il voto democratico, consentendo che l'ente Provincia diventasse un centro di collocamento per politici amici e non amici dei cittadini. Oggi le conseguenze più deleterie si hanno sul piano dell'edilizia pubblica, delle infrastrutture, delle strade e sempre più i territori si vanno depauperando, isolandosi completamente, in seguito all'incuria consentita dal rimpallo di responsabilità tra enti che fino a oggi i Governi hanno tollerato. Non possiamo più permettere che qualche amministratore, qualche tecnico e qualche "prenditore" di appalti, vantandosi di determinate cariche, vada ad infangare il buon operato del mondo della politica, dell'imprenditoria, degli ordini degli ordini professionali, con comportamenti non solo eticamente da condannare ma giuridicamente criminosi. In quest'ottica, questo provvedimento deve essere inteso come il trampolino di lancio di una vera e propria programmazione strategica e la maggioranza parlamentare che sostiene il Governo in carica interverrà con le misure di pianificazione pianificazione per semplificare anche le azioni di ristrutturazione, permettendo a cittadini e imprese di riprendere con serenità le proprie attività quotidiane per un effettivo miglioramento della qualità e della dignità della vita.

in queste prime settimane della XVIII legislatura, il decreto-legge n. 55 del 2018 è stato affrontato esclusivamente in sede di Commissione speciale, con particolare attenzione - un'attenzione quasi esclusiva - agli aspetti economico-tributari, che non esauriscono certamente i gravi problemi che hanno colpito le popolazioni interessate dal sisma. Non sarebbe stata possibile una soluzione alternativa, perché non esistevano le altre Commissioni, ma questo ha fatto sì che il documento cogliesse esclusivamente questa dimensione dei problemi e lo facesse secondo tre direttive molto precise: prima di tutto, la sospensione dei termini tributari e contributivi attraverso le ripetute proroghe, la possibilità di finanziamenti agevolati assistiti per il pagamento dei tributi sospesi e, in terzo luogo, questa sorta di rincorsa dei prolungamenti successivi, in cui lo Stato si offre di garantire il debito, ma né interviene per ridurre questo debito, né svolge un'azione positiva di risanamento rispetto alle ferite che il sisma ha prodotto. Peraltro, la cosa più ridicola è che la prima proroga, che cominciava il giorno del terremoto, sarebbe dovuta terminare sei mesi dopo. Ovviamente la tempistica italiana e l'esperienza di tutti gli altri terremoti dimostravano già che fissare termini in questo modo rappresenta un misto fritto tra ingenuità e incompetenza. Di fatto, dopo gli eventi sismici del 24 agosto 2016, che hanno colpito appunto Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, l'iniziale termine per la sospensione dei tributi è passato dal 16 dicembre 2016 al 30 novembre 2017, successivamente al 31 dicembre 2017 poi ulteriormente al 31 maggio 2018 e oggi, per quanto riguarda gli istituti autonomi per le case popolari situati nei territori colpiti dal sisma,

I primi a esprimere il fallimento di queste promesse sono proprio le popolazioni colpite dal sisma per i quali la pressione fiscale resta l'unica ottica attraverso la quale vengono letti i loro problemi. Possiamo Possiamo dire, di fatto, che mentre la pressione fiscale, sempre fin troppo pesante per tutti gli italiani, concedeva comunque un minimo di respiro puramente virtuale alle zone terremotate, le misure, che avrebbero dovuto facilitare la ricostruzione di case e strutture (comprese le scuole e gli uffici pubblici) e la ripresa delle attività lavorative (a cominciare da quelle produttive, ma con particolare attenzione anche all'area di servizi socio-sanitari), mostravano un rallentamento ai limiti dell'inerzia. Le strade sono visibilmente ancora occupate dalle macerie e dai detriti. La circolazione è fortemente limitata sia in termini di accesso che di velocità percorribile. Le case sono inagibili e per qualsiasi esigenza occorre spostarsi nei Comuni vicini non colpiti dal terremoto, aumentando la sperequazione che c'è tra chi ha sofferto per questa ferita e chi fortunatamente ne è stato esente. In altri termini, se le tasse dovute non sono altro che il prezzo pagato per ottenere servizi dallo Stato, qui a servizi a livello zero le tasse non le avrebbero dovute nemmeno pagare. I problemi sono affrontati nell'ottica di uno Stato creditore, che in modo pseudo magnanimo accetta di aspettare, ma non assume responsabilità concrete e tempestive per avviare la fase della ricostruzione. Pertanto, a due anni dal sisma, la vita appare ancora congelata in quelle zone in cui, peraltro, vige una burocrazia che rende assolutamente problematico procedere, sia pure con risorse proprie, alla ricostruzione e al rilancio di attività commerciali e imprenditoriali. Il ritorno a casa per la popolazione anziana, frastornata da spostamenti che equivalgono a sradicamenti di cui pagano un prezzo elevato anche in termini di salute con un aumento significativo delle patologie psicofisiche, è una delle tre richieste prevalenti. la rete sociale per i più giovani, a cominciare dalla scuola, ma includendo anche tutto l'insieme dei luoghi di incontro e di socializzazione; il lavoro per i giovani e meno giovani, obbligati ad abbandonare i loro territori per dare vita a una migrazione interna indispensabile per farsi carico delle proprie famiglie.

È mancata la percezione globale dei problemi delle popolazioni. Per questo è chiaro che non possiamo dare un voto positivo a questo decreto-legge. Probabilmente ci asterremo, ma la verità è che la tentazione di esprimere un voto negativo è di gran lunga maggiore.

2009, a L'Aquila e in Abruzzo: case, edifici, questura, prefettura, ospedale, la casa dello studente; la città di Onna completamente rasa al suolo, più di mille feriti, circa 65.000 sfollati, 309 vittime.

Marche il 26 ottobre e il 30 ottobre in Umbria, a Norcia, ore 7,40: il terremoto per intensità più forte del XXI secolo, circa 30.000 sfollati tra Marche e Umbria. Nel 2017, in Campania, due vittime. Sono dati e date che hanno segnato i nostri ultimi anni e che segnano anche i nostri ultimi giorni, e mettono a dura prova le nostre paure a causa della ininterrotta attività sismica che interessa la fascia tettonica alpino-appenninica. L'Italia è sempre in allerta e la politica deve essere sempre pronta e compatta. Dobbiamo essere sempre consapevoli e memori di tali eventi, coscienti ed imperterriti a risolverli quanto prima. Siamo obbligati a salvare sorrisi e speranze. Ovvio quindi che, come Lega, siamo favorevoli a che il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, con le dovute modifiche apportate di fretta, venga convertito in legge. Ringraziamo anche il Parlamento europeo, che ha stanziato 1,2 miliardi di euro dal Fondo di solidarietà europea per i 140 Comuni delle quattro Regioni interessate dal terremoto. L'utilizzo delle risorse, la scelta delle operazioni da eseguire e l'esecuzione delle attività di verifica e controllo sono state e sono di responsabilità dello Stato italiano, e voglio credere che le mani che hanno toccato questo denaro siano state mani responsabili e rispettose del dolore delle popolazioni terremotate. Presidente, onorevoli senatori, ho sempre creduto che, soprattutto in quest'Aula, ogni giorno è il giorno, ed oggi è il giorno per chiedere scusa per i ritardi, per le promesse non mantenute, per una burocrazia contorta e per la durezza della politica stessa, a volte. anche il giorno per rendere ancora onore ad un popolo sofferente; un abbraccio, perciò, che arrivi ai figli delle popolazioni terremotate, incolpevoli di vivere ancora in case di emergenza e crescere ancora senza certezze. Ma siate certi che, per la Lega, i loro figli sono i nostri figli; per la Lega, prima i terremotati; per la Lega, prima gli italiani.

questi pochi minuti che ho a disposizione, mettere in evidenza in quest'Aula una disparità di trattamento nel nostro Paese rispetto a calamita naturali che purtroppo si verificano. all'evento che, esattamente un anno dopo, il 21 agosto 2017, si è verificato nell'isola di Ischia e ha colpito alcuni Comuni di quest'isola. Ebbene, posso affermare senza timore di essere smentito

sintetizzo brevissimamente i danni che hanno riportato i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio il 21 agosto 2017 e che ad oggi non hanno trovato assolutamente risposta:

i posti di lavoro che si sono persi a causa dell'evento in maniera diretta sono 600, il calo delle presenze turistiche lo scorso anno, dopo qualche ora

e non solamente sui tre Comuni colpiti dal terremoto) un calo delle presenze turistiche che sfiora il 30 per cento. Sono dati ufficiali. Da parte

siamo ancora in regime di emergenza; non si intravede assolutamente un percorso di luce che possa far uscire dal *tunnel*

da un lato, a equiparare i Comuni danneggiati dell'isola d'Ischia agli altri Comuni dell'Italia centrale, stabilendo anche per i primi una serie di norme che agevolano e prorogano determinati tributi,

emendamenti che danno risposte e soluzioni a questi temi. Tantissime delle circa 2.000 abitazioni danneggiate in maniera irreparabile sono state costruite anni fa; su di esse pende istanza di sanatoria edilizia rispetto alle leggi dello Stato e non hanno avuto ancora concessione in sanatoria. Si tratta

passato. In Commissione, come diceva prima il Presidente nel suo intervento, si è lavorato senza demagogia con tutti i Gruppi, stabilendo questo pacchetto di emendamenti sarebbe stato ritirato per far sì che il Governo e gli uffici dei Ministeri avessero più tempo per poterlo esaminare in maniera compiuta e poter

Gruppo di Forza Italia, che i partiti, la maggioranza e il Governo sappiano rispettare gli impegni, sappiano analizzare e dare delle risposte certe a quelli che, come ho detto prima, sono i bisogni di comunità che vivono un momento di estrema difficoltà. Noi, come movimento politico, quando abbiamo avuto la responsabilità di guidare il Paese, abbiamo dimostrato che a a problemi normali si possono e si devono dare risposte normali ma che, rispetto a eventi straordinari, c'è bisogno di risposte straordinarie. Lo ha fatto il Governo del presidente Berlusconi, come si diceva prima, con il terremoto di L'Aquila. rubo solamente altri trenta secondi della vostra attenzione per dire che c'è anche un altro terremoto che potrebbe in maniera irreparabile

Una legge dello Stato che trova applicazione in tutto il territorio nazionale tranne che in Campania. Io invito i rappresentanti del Governo, invito i partiti che formano questa maggioranza di Governo, invito in modo particolare la Lega, che con noi ha condiviso il programma elettorale con il quale ci siamo presentati alle elezioni del 4 marzo, essere discontinui rispetto ai Governi del passato, anche rispetto ai Governi del centrodestra che non hanno saputo precedentemente dare una risposta compiuta a questo problema. Altrimenti, infatti, la Campania potrebbe trovarsi presto travolta da un nuovo terremoto.

Signor Presidente, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, membri del Governo, ci apprestiamo a convertire un decreto-legge in aiuto alle popolazioni colpite dai terremoti che nell'ultimo decennio hanno interessato la nostra penisola. Si tratta di un atto urgente che prevede prevalentemente proroghe a scadenze imminenti, scadenze che non possono maturare prima del superamento dello stato di emergenza. Il Centro Italia è ancora oggi soggetto a smottamenti, iniziati nove anni fa, in quella notte del 6 aprile che ha segnato la distruzione economica e sociale di un intero territorio, quello di L'Aquila e dei Comuni limitrofi. Vero è che la ricostruzione è partita, ma altrettanto vero è che essa procede a passi lenti, talmente lenti da far sentire quei cittadini soli ed abbandonati al loro dolore, dolore che rappresenta una grande ferita per l'Italia intera; dolore per la perdita di una parte del loro vissuto; dolore per la perdita di proprietà non ancora loro restituite; ferite aperte e che mai si rimargineranno per la perdita del bene più prezioso, quello dall'affetto dei propri cari venuti a mancare sotto un cumulo di macerie. trecento vittime e ottantamila sfollati avuti anche con il crollo di strutture pubbliche, come la casa dello studente e parti dell'ospedale e dell'università. Sento l'obbligo di menzionare in questa sede la distruzione dei sogni di ben 2.914 persone in Irpinia, nel lontano, ma non troppo, 1980. Il terremoto più devastante che ha comportato per la prima volta l'introduzione di interventi urgenti e dalla cui esperienza è nata l'imponente macchina della Protezione civile di cui oggi l'Italia è dotata. furono le vittime del sisma in Emilia-Romagna mentre se ne contano 299 nel più recente, che ha interessato le Regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Ogni qualvolta si verifica un tragico evento sismico, emerge una preoccupante impreparazione del Paese, nonostante siano note da tempo le criticità legate alle aree a maggior rischio. Oggi ereditiamo una drammatica condizione del patrimonio edilizio scolastico che, dai dati in nostro possesso e che verranno integrati al prossimo 31 agosto, per l'80 per cento non risulta adeguato alla normativa sismica vigente. Perché oggi Perché oggi ci troviamo a gestire una simile circostanza? Perché i nostri figli continuano a frequentare scuole insicure esponendo la loro vita a gravi rischi, come accadde a San Giuliano di Puglia? La ricostruzione è legata al palo: è inutile negarlo. Ci sono ancora tanti nodi burocratici da sciogliere per velocizzare i processi di ricostruzione, mentre le popolazioni interessate continuano a versare in condizioni di difficoltà economica e di sfiducia nei confronti delle istituzioni. Qualcosa è stato fatto, già, ma c'è ancora molto da fare e bisogna capire dove è fondamentale intervenire per essere davvero risolutivi, evitare sperperi e indirizzare il denaro pubblico verso la

Commissione speciale, alla quale è stato assegnato l'urgente disegno di legge n. 435, è stato purtroppo impossibile affrontare accuratamente tutte le problematiche e poter proporre emendamenti al decreto-legge, per migliorare le attuali condizioni in cui si trovano i cittadini terremotati. La decisione presa dal commissario straordinario di chiudere gli uffici territoriali per la ricostruzione - ad esempio - produrrà - a mio avviso - un allungamento delle tempistiche nell'istruzione delle pratiche, sottraendo un importante servizio di prossimità territoriale a tutti gli attori impegnati nella ricostruzione. Mi auguro che il lavoro svolto in Commissione speciale riceva l'approvazione di voi tutti, colleghi, con la consapevolezza che il nostro lavoro non termina qui: sarà necessario tornare a breve sulla spinosa tematica con proposte finalizzate alla rimozione di quei blocchi troppo troppo spesso di carattere burocratico e politico. L'Italia è un Paese altamente sismico a causa della sua posizione lungo il margine fra due placche tettoniche in movimento, quella eurasiatica e quella africana. È arrivato il tempo di agire sulla prevenzione e non sull'emergenza, com'è stato sempre fatto fino ad ora. È assodato che gli interventi fatti senza una programmazione puntuale sono costati cifre enormi e non hanno non hanno evitato tragedie che diversamente, con l'intervento preventivo sulle note criticità del nostro territorio, sarebbero state evitate. Bisogna entrare nell'ottica che ci troviamo sì, in una situazione post-sisma, ma la realtà dei fatti è che siamo tutti chiamati a valutare e risolvere la situazione di allarme sotto il faro illuminante della prevenzione. Questo è il Governo del cambiamento e cambieremo il modo di affrontare il problema e di fare politica.

onorevoli colleghi, il primo dato che ci viene da sottolineare in questa discussione sul decreto-legge riguardante il terremoto fa

Ebbene, nel giro di pochi mesi - tra i sei e i nove - la gran parte delle persone che era stata sfollata dalle proprie case è rientrata non in casette fatiscenti o che si è dovuta costruire, aspettando e litigando con le amministrazioni che sono andate naturalmente e burocraticamente a contestare gli abusi (vedi la vicenda di nonna Peppina che stiamo risolvendo oggi), ma dentro delle case vere.

con la generosità della Provincia di Trento solo una o due rimangono abitate da famiglie che erano state sfollate; nel frattempo stanno tutti rientrando nelle proprie case, che stanno ricostruendo. Oggi, quel patrimonio edilizio non è un problema per l'amministrazione e per il Comune, ma è anzi una risorsa. Quelle case infatti sono state abitate da giovani e da nuove famiglie e quindi un paesino di 300 o 400 abitanti, che si andava spopolando, come tante aree interne della nostra Nazione, è tornato ad avere una crescita demografica e con le entrate dell'affitto, delle locazioni di quelle casette, oggi tiene l'IMU, la TASI e la TARI al minimo possibile, agevolando quindi la vita dei cittadini. Oggi abbiamo invece sotto gli occhi cosa accade quando un altro Governo si è trovato ad affrontare i terremoti avvenuti negli ultimi anni. Il fatto che siamo qui, in Aula, a votare delle proroghe di scadenze, o a prorogare la vigenza dello stato di emergenza, denota già il fallimento di quel Governo e del metodo di gestione dell'emergenza e della straordinarietà eventi. Quando lo Stato interviene su una vicenda del genere e stabilisce un tempo congruo entro il quale bisogna dare delle risposte - quindi su quel tempo misura la sospensione dei pagamenti, lo stato di emergenza per le procedure più accelerate e più straordinarie e così via - e poi si avvicina regolarmente quella scadenza e si rende conto che è ancora tutto drammaticamente fermo, per cui c'è bisogno di tornare in Parlamento e fare delle proroghe, di sei mesi

perversa, che credo sia necessario evidenziare. Pongo a tutto il Parlamento un problema: si è smantellata la Protezione civile come organo deputato ad affrontare le emergenze, dando la stura a una polemica speciosa, che

smantellando la Protezione civile, ma semmai smettendo di affidarle operazioni per eventi che non rientravano nell'emergenza e nella straordinarietà. Quando però si verifica

al di là delle persone coinvolte, tutte dignitose e tutte sicuramente meritevoli della nostra stima personale, da Errani fino a De Micheli. Non stiamo discutendo le

scarse e sbagliate che gli sono state messe a disposizione, nel modo in cui si è frammentato il processo decisionale fra quattro Regioni, con commissari che si sono relazionati con quattro uffici diversi, Regione per Regione. E ciò è accaduto perché bisognava uccidere la Protezione civile civile e smantellare un buon lavoro, un buon esempio di amministrazione, capace di affrontare l'emergenza; un sistema che ci invidiava il mondo intero e rispetto al quale abbiamo invece fatto un disastro, cedendo a logiche e polemiche pretestuose. E a quelle polemiche ne è seguita un'altra

E figuriamoci che baffo si farà degli ordini del giorno che siamo stati invitati a presentare e sottoscrivere in cambio del ritiro degli emendamenti. Voglio dire una cosa ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che, per cinque anni, hanno fatto un'opposizione dura e pesante nei confronti del Governo

Eventuali subemendamenti potranno essere presentati entro le ore 20 di questa sera, affinché la Commissione bilancio possa esaminarli fin dalla seduta di domani mattina. È iscritto a parlare il senatore Astorre. Ne ha facoltà. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il provvedimento in esame, adottato dal precedente Esecutivo, sono state affrontate le più urgenti problematiche, intervenendo - da un lato - sul regime sospensivo, con l'allungamento della durata delle proroghe per gli adempimenti amministrativi più importanti e onerosi per cittadini, imprese e Comuni coinvolti, - dall'altro lato - sulla semplificazione amministrativa, finalizzata a rendere più celere il processo di ricostruzione del patrimonio abitativo e infrastrutturale. Voglio dire che non si può non apprezzare la vicinanza, mostrata con la visita del presidente del Consiglio Conte, lo scorso 11 giugno, ad alcuni Comuni colpiti dal sisma, quali Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Tuttavia, la vaghezza e la genericità con le quali questo Governo si è approcciato al *Dharma* generale degli eventi sismici, sia nel corso delle dichiarazioni programmatiche, in cui si è fatto solamente un brevissimo cenno al sisma (esclusivamente per annunciare una imminente visita del Governo), sia nel cosiddetto contratto di Governo, lasciano sul terreno forti preoccupazioni. Avrei preferito, avremmo preferito che il Governo si fosse presentato in Aula, nel corso della fiducia, declinando in maniera dettagliata le iniziative e i provvedimenti che intende adottare, con la rapidità e l'urgenza che un simile dramma richiede. Non va infatti dimenticato che il provvedimento che stiamo per licenziare porta la firma del precedente Governo. Ricordare questo aspetto è importante, e non tanto per rivendicarne la paternità, quanto per rilevare, con grande preoccupazione, l'assenza di un'attenzione politica verso una delle più impellenti priorità del nostro Paese. Non sappiamo come questo Governo e la sua maggioranza intendano rilanciare, con impulso ancora maggiore, la fabbrica di quei territori, ovvero il sistema agroalimentare, il sistema dei parchi, il sistema ambientale, il sistema produttivo legato alla terra e all'ambiente. Non conosciamo qual è l'ispirazione di fondo che animerà il processo di ricostruzione del tessuto umano e relazionale di quelle comunità, caratterizzate da una straordinaria ricchezza di storia e di eccellenze culturali. quali saranno gli interventi che si intendono adottare, in via strutturale e non emergenziale, al fine di impedire quel processo di dispersione e di fragilità demografica che accomuna purtroppo moltissime aree interne delle nostre Regioni italiane? Si tratta di un processo che, pur non essendo attribuibile a questo o al precedente Governo, non può non trovare il suo legittimo spazio all'interno del programma politico di un Governo appena insediato. Al contrario, sarebbe stato molto apprezzato, soprattutto dalle popolazioni ancora traumatizzate da quegli eventi terribili, se da un neonato Governo fosse stata indicata una rotta, una strategia per provare a rallentare, a trattenere, a invertire quel processo di impoverimento demografico. Ebbene, tutto ciò non lo conosciamo, perché, al di là di qualche annuncio propagandistico che può andare bene per i *social*, ma non certo per la vita concreta delle persone che soffrono, questo Governo e questa maggioranza non hanno ancora espresso con chiarezza e decisione i loro intendimenti politici e programmatici sul tema. Alla piaga del terremoto, che purtroppo con eccessiva frequenza ci ricorda quanto sia fragile e instabile il nostro territorio e quanto sia elevata la sua esposizione al rischio sismico, come pure ai rischi di dissesto idrogeologico, frane e alluvioni, si affianca un fenomeno di carattere sociale fatto di comportamenti scorretti e disonesti e di azioni fraudolente, che, approfittando di situazioni di emergenza e di abbattimento morale, tenta di ottenere indubbi benefici di natura economica, e non solo. Quanto è emerso alcuni giorni fa da un'indagine della Guardia di finanza di Camerino è inquietante: in una nota della Guardia di finanza si parla di 120 casi, per un totale 500.000 euro, mentre i sequestri già eseguiti non è una novità: in passato, in simili situazioni, si sono verificati gli stessi fatti. È vero che è ancora tutto da dimostrare e che vale sempre e per tutti la presunzione di innocenza. da chi ha la responsabilità di governare il Paese ci aspettavamo almeno una parola di denuncia di un malcostume che, lucrando sul dolore di intere comunità, sottrae risorse di cui avrebbero estremo bisogno coloro che, a causa di un evento drammatico, hanno perso tutto: i familiari bisogno coloro che, a causa di un evento drammatico, hanno perso tutto: i familiari e i frutti dei sacrifici di una vita. Bastava una parola per affermare che l'Italia è altro, che l'Italia è il Paese della solidarietà, dell'aiuto reciproco, della cooperazione e della convivenza porta a porta. L'Italia è il Paese dei borghi, proprio come quelli che sono stati colpiti da quei terremoti, nati e cresciuti con case adiacenti, che dipendono l'una dall'altra, in maniera solidale, perché il muro dell'una e il muro dell'altra quasi si parlano.

approvato identico a quello emanato dal precedente Governo, ma che rispondesse a esigenze concrete delle comunità colpite dagli eventi sismici. Questa è stata la prima scelta che abbiamo avuto di fronte. Potevamo considerare questo l'ultimo decreto-legge del Governo Gentiloni Silveri o trasformarlo, cambiandolo, nel primo decreto-legge del Governo Conte. Sapevamo quali sarebbero stati i problemi, dettati dalla situazione di un Governo appena insediato, dai limitati tempi e dalle limitate risorse a disposizione. Sapevamo che non sarebbe stato un atto perfetto, ma sapevamo altresì che sarebbe stato un atto migliore. Di fronte a questo, la nostra è stata una scelta obbligata, è stata una scelta obbligata, perché il Governo del cambiamento è del cambiamento se è in grado di dare, sempre e comunque, le risposte che può fornire, nelle condizioni date. E questa è la scelta che abbiamo voluto voluto compiere. Mi rivolgo a chi ha ironizzato sul contratto, a chi ha ironizzato sul saluto e sul pensiero conclusivo del presidente del Consiglio Conte al termine del suo intervento in quest'Aula, che ha ricordato proprio le popolazioni colpite dal terremoto. rivolgo a chi ha ironizzato sulla visita nelle zone colpite dal terremoto e soprattutto ai senatori Astorre e D'Alfonso, che sembrano oggi arrivati qua da Marte. rivolgo al senatore presidente D'Alfonso, perché è doppiamente spudorato quando parla di ipocrisia, di immoralità e si appella all'onestà intellettuale. Con quale coraggio si può parlare di onestà intellettuale quando si chiede conto a un Governo che è in carica da meno di due mesi e si è rappresentanti di un partito che ha sostenuto un Esecutivo che in quasi due anni non ha dato risposte alle popolazioni colpite dal terremoto? Ovviamente è in buona compagnia. Noi condividiamo la preoccupazione dei senatori del PD e il loro comunicato stampa; anche noi pensiamo che non si possa andare nelle zone terremotate a fare le passerelle. Il problema è che è quanto hanno fatto loro per mesi, lasciando a noi Gruppi L-SP e M5S)*. Ma su questo tornerò fra poco. Devo dire che sicuramente è stato più onesto intellettualmente il senatore Grimani. Ma, forse, D'Alfonso e Grimani non si sono parlati. Forse D'Alfonso era in Abruzzo a fare il Presidente.

Il quadro emerso dalle audizioni che abbiamo comunque voluto svolgere, nonostante i tempi ristretti, chiamando tutti, dalle Regioni ai Comuni, dalle associazioni di categoria ai professionisti, passando per i comitati dei cittadini,

«Vediamo come stanno le cose, confrontiamoci, risolviamo i problemi, colmiamo le lacune, correggiamo gli errori». C'è stata la presunzione di avere la verità in tasca e di andare avanti negando i problemi concreti che le persone vivevano nelle zone terremotate tutti i giorni. Ebbene, sarà poco quello che è stato aggiunto al momento in Commissione speciale, e che troverà conferma qui in Assemblea. È poco forse per chi non vive le situazioni che ci ricordava prima il collega Pazzaglini. Per le persone coinvolte, però, non è Sapere che la propria pratica, che giaceva fra i condoni pendenti, può finalmente andare avanti; che la ricostruzione della propria vita, oltre che della propria casa, può prendere il via, è tantissimo per quelle persone.

un'esperienza che penso non abbia eguali per quanto possa essere terribile. Si potrebbe tornare, allora, sugli altri emendamenti approvati; ne cito soltanto uno per dare la misura di quanto sia stata alla ricostruzione. Possibile che nessuno abbia pensato che un Comune terremotato, con il 90 per cento degli edifici distrutti, debba essere esentato dalle penali per il mancato raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata? A distanza di mesi avevamo la vergogna di cittadini che dovevano pagare, con la

È stata criticata - dicevo prima - la passerella, la visita del *premier* Conte nelle zone colpite dal terremoto probabilmente lo sarà anche quella del Ministro dei beni culturali che era lì oggi - come ha ricordato il collega Lucidi - insieme al Sottosegretario all'interno. Noi, però, visitiamo le zone colpite dal terremoto normalmente il giorno dopo aver risolto i problemi, perché è di ieri la firma, da parte del Ministro dell'interno, dell'atto che sblocca 9,7 milioni di euro di straordinari arretrati dei Vigili del fuoco.

il collega Pazzaglini ha ricordato la deportazione - per così dire - delle popolazioni che per mesi hanno vissuto negli alberghi (dovevano starci poche settimane). Io ho avuto la fortuna - e dico la fortuna - di abitare nel Comune di Passignano sul Trasimeno che ha accolto decine di sfollati del terremoto. Con loro abbiamo condiviso le feste dei figli; abbiamo condiviso la messa in parrocchia; abbiamo condiviso gli incontri.

Il sisma che ha sconvolto la mia Regione e il centro Italia è stato infatti - inutile dirlo - devastante, anche in considerazione del fatto che è arrivato in una Regione già terribilmente colpita dal terremoto del 2009. In aggiunta a ciò, il territorio montuoso che caratterizza l'Abruzzo, coniugato con il maltempo dello scorso inverno, ha contribuito a peggiorare una situazione già estremamente precaria.

Ebbene, a fronte di tutto ciò, ci si sarebbe aspettati dal Governo precedente una particolare attenzione verso le popolazioni colpite. Invece, mi duole sottolineare come la gestione del sisma sia stata confusionaria, caotica e a tratti irragionevole. In situazioni tragiche come queste è innegabile che occorra mettere da parte in un primo momento la polemica politica e lasciare che i Governi si occupino di fronteggiare l'emergenza, e così è stato fatto. Non abbiamo minimamente fatto polemica ma, in un secondo momento, è altrettanto vero che è apparso in modo evidente l'enorme divario tra la gestione dell'evento sismico da parte del Governo Berlusconi del 2009 rispetto a quella inadeguata e successiva del Governo Gentiloni Venendo al decreto-legge in esame, noterete come il versamento dei tributi - ad esempio - sia stato solo sospeso. Al contrario, il Governo Berlusconi aveva provveduto a ridurre in modo estremamente significativo il contributo fiscale dovuto per le popolazioni colpite dal sisma. Non solo: il decreto-legge in discussione prevede una rateizzazione del totale dovuto non sufficientemente diluita nel tempo. In merito ho presentato, come primo firmatario, un emendamento che ricalcava esattamente le misure prese dal Governo Berlusconi in occasione del sisma del 2009 a L'Aquila. Ho chiesto sostanzialmente che il contributo IRPEF fosse ridotto del 60 per cento e che le rate fossero portate da 60 a 120: stesso identico trattamento che ebbero gli aquilani nel 2009. Ebbene, tale emendamento è stato respinto dal Governo in carica i cui esponenti, in campagna elettorale, hanno criticato duramente la gestione del terremoto da parte del Governo Gentiloni Silveri e lo hanno fatto anche oggi, qui in Aula. Eppure, quando è arrivato il momento di intervenire nel concreto per portare sollievo a una popolazione stremata, a persone che hanno perso tutto, esattamente come chi avevano tanto criticato. Evidentemente in questo Paese ci sono terremotati di serie A, quelli che sono stati trattati da Berlusconi nel 2009, e terremotati di serie B, quelli del terremoto del 2016-2017, maltrattati dal Governo precedente e da quello attuale. Sono curioso di capire, a questo punto, cosa ne sarà degli altri emendamenti presentati. Ci sono Comuni come Catignano, Civitella Casanova, Penne, Penna Sant'Andrea e Basciano in Abruzzo irragionevolmente esclusi dal cratere; Comuni che hanno subito danni dal sisma sia concretamente che collateralmente; Comuni che hanno dovuto fronteggiare anche l'emergenza neve dello scorso inverno in un territorio già stremato dal terremoto. La città di Penne - per esempio pare sia vittima di quello che non mi faccio problemi a definire come un vero e proprio accanimento: a quanto pare, il Governo Gentiloni Silveri ha voluto fingere che questo Comune non sia stato colpito dal sisma; ha poi cancellato con un colpo di spugna il fatto che sia stata proprio l'amministrazione di Penne a prestare i soccorsi nella tragedia di Rigopiano. Non contenti, hanno deciso anche di non sospendere i piani sanitari che prevedono la chiusura di strutture ospedaliere fra cui proprio quella di Penne. L'ospedale di questo Comune è stato fondamentale nella tragedia di Rigopiano e non solo: raccoglie un bacino d'utenza di 60.000 persone che sarebbero, in caso di chiusura, costrette a dirigersi verso l'ospedale di Pescara. Sapete quanto ci vuole da Penne in provincia di Pescara ad arrivare a Pescara? Occorre quasi un'ora di auto e questo creerebbe un disagio enorme. Ebbene, ho presentato un ulteriore l'emendamento per scongiurare quello che sarebbe un ulteriore schiaffo alla popolazione di quei territori. I due emendamenti sono stati invece, purtroppo, trasformati in ordini del giorno, cioè aria fresca. Questa è la verità. In Commissione speciale mi è stato chiesto - il mio senso di responsabilità ha fatto sì che io comunque accettassi - questa secondaria strada, ma non è molto: in realtà, è veramente molto poco. Mi auguro che questo Governo non si limiti - come ha fatto finora - a stigmatizzare, quando era all'opposizione, la gestione a marchio PD per poi confermarne invece le misure prese, ma se ne discosti con i fatti, dando un contributo effettivo ai Comuni dimenticati dal precedente Esecutivo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Mi chiedo, altresì, a cosa sia servito esattamente ascoltare i sindaci: sono venuti in Commissione speciale e hanno parlato; non voglio pensare che la loro audizione sia stato un atto dovuto o peggio ancora di propaganda. L'Esecutivo ha il compito e il dovere di dimostrare davanti a tutto il Paese che davvero, al di là degli *slogan*, certi italiani bisognosi vengono prima degli altri. Alla prova dei fatti, mi sembra che non sia così; anzi, mi sembra che la gestione del sisma da parte del Governo gialloverde sia speculare e si muova nel solco della gestione a targa PD, visto che - ci tengo a ribadirlo - è stato bocciato un emendamento che prevedeva la riduzione dell'IRPEF per le popolazioni colpite. Non cadiamo nell'errore di considerare tale questione solo in termini numerici ed economici: il problema prima ancora che legale e sociale è culturale. La gente si aspetta dallo Stato che mostri la benevolenza di un padre e non che si manifesti come una severa matrigna. Le zone terremotate hanno bisogno non solo dell'aiuto materiale per risorgere, ma anche di una particolare sensibilità istituzionale affinché non si disperda quel patrimonio immateriale fatto di persone che vivono e operano in un contesto sociale di cui fanno parte e di cui sono l'identità. Se davvero questo Governo vuole fare la differenza, deve ascoltare la voce dei cittadini e di chi davvero conosce e vive quei territori ogni giorno. giorno. Da parte mia non mi arrenderò. Non lascerò sulle spalle delle popolazioni colpite un carico di tributi iniquo, in considerazione di ciò che hanno passato e, quindi, sono stati ripresentati anche gli emendamenti bocciati in Commissione. Questo Governo dovrà dire a me, all'Assemblea e soprattutto alle popolazioni colpite che non meritano un trattamento speciale, che tutto ciò che hanno subito non vale una riduzione del carico fiscale.

che si sono manifestati in aree che ho investigato personalmente e nelle quali risiedo. È facile rendersi conto come in tutta la Penisola italiana sia grande il rischio sismico: terremoti in aree considerate a rischio basso o nullo come l'Emilia-Romagna rivelano come nessun settore della Penisola sia scevro da pericolosità. Le aree più pericolose sono ben note da tempo e in genere sono rappresentate da fasce di dislocazioni lineari allungate. Durante i terremoti, però, la sollecitazione mobilizza o rimobilizza le aree interessate da dissesto, in particolare le aree franose, che in alcuni settori della Penisola ricoprono oltre il 70 per cento del territorio. In tali aree si dovrebbe evitare di intervenire o farlo solamente se non ci sono alternative e, in tal caso, farlo con le dovute precauzioni e gli accorgimenti tecnici. Ci sono inoltre criticità legate a motivi storico-architettonici dato che le nostre magnifiche città sono state edificate in periodi in cui le tecniche costruttive non tenevano conto dell'esigenza di una progettazione antisismica. Mi fa piacere che questo decreto-legge venga emanato con l'avallo di tutte le forze politiche. È questo lo spirito che dovrebbe guidare l'approccio a un problema trasversale e immanente. Il decreto-legge ha avuto dei vincoli a cui la maggioranza attuale ha dovuto adeguarsi. È nato come una proroga di scadenze per il supporto ai territori che, a due anni di distanza dagli eventi, sono ancora in condizioni emergenziali. I membri della Commissione, indipendentemente dagli schieramenti politici, hanno presentato emendamenti migliorativi che il Governo, pur se appena insediato, ha fatto il possibile per accettare. Abbiamo ancora molto da fare per impedire che eventi di questa tipologia arrechino danni e, soprattutto, lutti ai nostri territori. È molto difficile e, soprattutto, costoso mettere in sicurezza i centri storici. Le nostre edificazioni dovrebbero essere realizzate con norme antisismiche in modo che, come avviene in una Nazione come il Giappone, superino con minori danni e vittime terremoti di magnitudo ben più elevata di quella che ha colpito il nostro territorio. Stupisce, infatti, che nell'area del cratere siano collassate strutture realizzate quando nella zona erano già in vigore normative antisismiche. Su queste questioni sta comunque indagando la magistratura e spero che chi, come il sottoscritto,

a seguito del terremoto e vi assicuro che vedere i volti di persone, in particolare di bambini, rimasti uccisi dal crollo delle proprie abitazioni, è veramente straziante. Il nostro territorio è a rischio, talora a rischio veramente elevato. È necessario recuperare il tempo perduto per la conoscenza approfondita del territorio dato che la cartografia geologica ha uno stato di attuazione talora scarso e, comunque, estremamente variabile da Regione a Regione. Talora la frammentazione normativa ha condotto ad avere prodotti diversi tra Regioni limitrofe e purtroppo saranno necessari interventi per uniformarli. Mentre in molti Stati europei il servizio geologico ha una regia Nazionale nel nostro Paese La microzonazione sismica, che permette di limitare le aree più critiche, è nota solo per un numero limitato di Comuni. A seguito dell'evento, nell'area del cratere è stato fatto uno sforzo elevato per produrre la microzonazione sismica di terzo livello per le zone dove è stata indirizzata la ricostruzione, anche se purtroppo l'esiguità delle cifre messe a disposizione ha impedito di ottenere dati esaustivi. Questo strumento avrebbe dovuto essere utilizzato in tutti i nuovi piani strutturali e per le nuove edificazioni. Ho sentito in quest'Aula richiamare ancora la necessità di costruire un ponte sullo Stretto di Messina. Ricordo a tutti che la pericolosità sismica di una Regione è calibrata sul massimo terremoto noto che nell'area dello stretto è di magnitudo di poco superiore a 7. Nessuno può, però, assicurare che nell'area non si possa manifestare un terremoto con magnitudo anche superiore e, purtroppo, molte evidenze geologiche, anche in altre Regioni italiane, suggeriscono che tali eventi sono stati e possono ripetersi. I costi della realizzazione del ponte salirebbero ulteriormente rispetto ai preventivi attuali. Nell'ambito di una programmazione con un territorio nazionale pieno di problemi che richiederanno ingenti impegni economici è saggio concentrarsi sulle priorità che garantiscono investimenti su settori strategici. Sembra inutile spendere denaro sul ponte quando poi il resto d'Italia necessita di un ulteriore massiccio piano di investimenti per la sistemazione delle strade e delle scuole. Credo che tutti congiuntamente troveremo il modo di superare i problemi legati alle lievi difformità che finora hanno impedito l'inizio della ricostruzione. Non dobbiamo dimenticare che la maggior parte delle persone hanno perso le proprie realtà insediative che vivono in piccoli moduli abitativi e che larga parte del tessuto produttivo è stato distrutto o compromesso. L'aspetto psicologico gioca un ruolo importante nella ricostruzione che tutti auspichiamo. Ancora oggi, per raggiungere alcuni importanti settori dei crateri sono necessarie ore

essere uniti e senza sciacallaggi di sorta. Siamo e rimarremo uniti e vicini alla popolazione in tutti i modi possibili, e assicuriamo che questo decreto-legge non esaurirà il nostro mandato al passaggio fra due legislature. Vi ringrazio per l'attenzione.

Signor Presidente, ho ascoltato con interesse e ringrazio tutti i colleghi intervenuti che hanno dato un contributo anche alla discussione generale su questo disegno di legge di conversione del decreto-legge,

ciclicamente, vede abbattere sul proprio territorio. Questo è vero: non tutti gli strumenti usati dopo un evento catastrofico sono stati riutilizzati in un altro. Questo ci dà il segnale di una mancanza, forse quella di - chiamiamolo così - un piano generale di gestione delle emergenze che abbia uno scheletro comune di tutti quelle misure, anche in termini di aiuti fiscali e di agevolazione alle imprese o di procedure per la ricostruzione, e anche di procedure di intervento sull' emergenza stessa. La casetta, i prefabbricati, le SAE: ogni volta c'è questo dibattito. È vero che ogni territorio probabilmente ha delle esigenze proprie, legate alle specificità di quell'area. Ma io ritengo che il Parlamento debba fare uno sforzo per capire se sia possibile avere un ossatura, uno schema che ci consenta di intervenire in modo immediato, rapido, consapevole, con gli stessi strumenti, per dare risposta a tutte le persone colpite da eventi calamitosi. Deve farlo in una

L'operazione che questa maggioranza, assieme al Governo, ha cercato di fare si riassume sostanzialmente

L'abbiamo fatto perché in questo modo, ragionando sulla legge di bilancio, molte delle previsioni che erano in scadenza anche prima di quella data (che non abbiamo prorogato esclusivamente per poterlo con maggiore certezza e con maggior impatto dal 2018 in poi), le potremo fare sulla legge di bilancio. Sarà quella l'occasione in cui daremo le risposte che molti colleghi oggi hanno chiesto. Non c'è nessuna norma agevolativa che andrà in scadenza prima del 31 dicembre 2018. Abbiamo allineato anche la scadenza dello stato d'emergenza, ossia il momento in cui termina lo Stato d'emergenza, con quello in cui termina la struttura commissariale. Da questo punto di vista, permettetemi di dire che nei giorni scorsi ho letto diversi articoli di quotidiani,

Tale struttura è viva al momento, fino al 31 dicembre 2018. C'è già un ordine del giorno, che è stato ovviamente accolto, perché è evidente che la struttura commissariale non morirà al 31 dicembre 2018.

volendo ovviamente allineare la scadenza della gestione d'emergenza con la proroga della struttura commissariale (avendolo fatto fino al 31 dicembre 2018), prorogare anche la struttura commissariale avrebbe

al collega Saccone che prima ha detto che dovrei essere in imbarazzo perché all'interno del provvedimento in discussione non c'è nulla. Io credo che lo abbia detto in un modo non negativo e polemico, nel senso che posso comprendere il ruolo dell'opposizione. Io invece mi sento orgoglioso di aver potuto contribuire, con le mie piccole capacità tecniche e ancora più limitate capacità politiche, a tenere assieme questo decreto-legge e le modifiche che stiamo apportando, coinvolgendo una maggioranza

ma che devono semplicemente risolvere i problemi di quei disgraziati cittadini che si sono trovati senza casa, senza lavoro e senza prospettive. *(Applausi dai Gruppi di aver potuto contribuire a dimostrare che non ci si può dividere. Ringrazio quindi tutti i colleghi che hanno interpretato questo mio spirito e che oggi hanno svolto degli interventi riconoscendo il nostro lavoro. Io credo che ci aspetti una serie di votazioni su diversi emendamenti; molte cose le abbiamo dette e le affronteremo. L'ultima cosa di cui mi sento orgoglioso - lo dico - lo dico sinceramente - è quella di aver potuto mantenere un impegno che avevo preso in quest'Aula con tutto il Senato: mi riferisco a quello di capire se c'era la possibilità di intervenire già oggi, attraverso un emendamento del relatore, sulle piccole difformità edilizie che stanno bloccando molte parti della ricostruzione. Oggi ho depositato questo emendamento dopo un lavoro che - ve lo assicuro - è stato faticoso, ma grazie al contributo di tanti siamo riusciti a predisporre un testo che tenga insieme la necessità di ripartire con la ricostruzione con quella di non aprire eccessivamente le maglie a interventi che non erano leciti. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP).* Noi abbiamo fatto questo lavoro e sono orgoglioso di averlo potuto presentare come emendamento del relatore.

Signor Presidente, colleghi, ho chiesto di intervenire per ricordare in Aula il collega Mario Santi, senatore della Repubblica dal 1972 al 1979, eletto nella VI e nella VII legislatura nelle liste della Democrazia Cristiana. Nato a Lucca ma vissuto a Prato, Mario Santi è venuto a mancare a novantaquattro anni sabato 23 giugno, nella sua casa e nella sua città, circondato dai suoi familiari. Da quel momento fino ai funerali, che si sono celebrati lunedì in cattedrale, praticamente l'intera città di Prato, senza distinzioni politiche, si è stretta attorno alla famiglia manifestando nei confronti del senatore Santi stima, gratitudine e affetto. Docente di filosofia al liceo Cicognini di Prato, fortemente impegnato nel servizio alla comunità pratese in ruoli amministrativi di rilievo, Mario Santi è stato attivo protagonista nel movimento cattolico. Era legato a La Pira e si sentiva vicino alle posizioni politiche del sindaco di Firenze. In Senato, Santi è stato nella VI legislatura membro delle Commissioni affari costituzionali e lavori pubblici, poi nella VII legislatura della Commissione affari esteri e della Commissione consultiva per i regolamenti CEE. In entrambe le legislature ha fatto parte della Commissione speciale per i problemi ecologici. Il suo impegno parlamentare si è incrociato con gli anni più drammatici del nostro Paese, culminati nella tragedia del rapimento e dell'assassinio del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. L'ultima uscita pubblica di Mario Santi è stata qualche settimana fa per un incontro dedicato proprio al quarantesimo della morte di Moro, quasi a sigillo del segno doloroso che quella tragedia ha lasciato in modo indelebile su lui, professore come Moro, che conosceva e stimava, come su una intera generazione di democratici cristiani e su tutti coloro che l'hanno vissuta e subita. Stimato dai colleghi di tutti i Gruppi, Mario Santi nel suo lavoro parlamentare si è fatto apprezzare per un'attività legislativa in cui non mancava mai una dimensione di umanità e di grande cultura. Credo sia giusto, e so di interpretare il sentimento di tutti i colleghi, che l'Aula del Senato gli dedichi un omaggio ed un ricordo insieme alla gratitudine per l'impegno e la passione civile che ha profuso nel suo ruolo di senatore. Alla moglie Anna, alle figlie e ai figli, Ilaria, Francesco, Domenico, Tommaso e Caterina, che gli sono stati amorevolmente vicino fino all'ultimo le più sentite condoglianze e il senso di partecipazione al loro dolore.

onorevoli colleghi, distratti membri del Governo, nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 giugno si è verificato un nubifragio nella provincia di Vibo Valentia, in particolare nei comune di Nicotera a Joppolo. Le piogge torrenziali che hanno colpito queste zone hanno provocato fiumi di fango e detriti che, a loro volta, hanno provocato l'evacuazione di molte aree di questi due Comuni. A Nicotera è ceduta un'abitazione, fortunatamente disabitata, e in altre zone hanno ceduto i muri di contenimento. Nel quartiere chiamato Marina, invece, gli abitanti sono stati costretti a lasciare le loro case per paura dell'esondazione di un fiume. La rete telefonica fissa è saltata e il traffico ferroviario ha subito diversi rallentamenti. A Joppolo la situazione non è stata diversa, con danni e disagi diffusi su tutto il territorio comunale. Senza contare il fatto che sono caduti i muri e che solo per un caso fortuito non ci sono state vittime.

Questo è grosso modo lo scenario relativo agli effetti del violento nubifragio del 17 e 18 giugno. Naturalmente, non è ancora possibile fare una stima precisa dei danni nelle due cittadine e nell'intera provincia di Vibo Valentia. I due Consigli comunali, nel frattempo, hanno chiesto formalmente la dichiarazione dello stato di calamità naturale. Una dichiarazione che, dal mio punto di vista, deve essere assolutamente accolta affinché le popolazioni colpite possano far fronte agli ingenti danni provocati dal nubifragio e sentano forte la presenza dello Stato. Tengo a ricordare che la Provincia di Vibo Valentia purtroppo non è nuova ad episodi del genere, come dimostrato dalle tremende alluvioni verificatesi non molti anni fa. Per questo ritengo che il Governo debba fare tutto il possibile, e naturalmente con estrema celerità, per dare risposte concrete ad un territorio fragile e ad una popolazione che ha il diritto di vivere in perfetta sicurezza all'interno delle proprie abitazioni e del proprio territorio comunale. *(Applausi dal

link apre una nuova finestra") su un fatto che ritengo rilevante e che sta assumendo contorni inquietanti, perlomeno per quanto si può apprendere da ciò che dell'inchiesta giudiziaria cui mi riferisco stanno scrivendo i giornali: sto del fatto che non sono stati trovati sui conti di un primario partito di Governo i denari

al Ministro della giustizia il 17 aprile scorso e, se era comprensibile la mancanza di risposte nelle more della formazione di un Governo, non sono più comprensibili silenzi, meline meline e fughe dal dovere di dare chiarimenti ora che un Governo c'è; dunque questo fatto necessita chiarezza nel più breve tempo possibile. Ho chiesto al Ministro della giustizia di dirci che cosa sa di questi fatti, quali valutazioni gli ispirano e quali azioni intende eventualmente adottare in merito a queste circostanze che, ripeto, sono allarmanti ed inquietanti, oggettivamente e per almeno altre due ragioni. La prima è che riguardano un primario partito di Governo e il suo rapporto di correttezza nei confronti dello Stato; la seconda è che per il suo ruolo di capo politico di quel movimento è il Ministro dell'interno in prima persona che dovrebbe sentire la necessità e il dovere istituzionale, per il ruolo che ricopre, di uscire da qualsiasi mutismo, da qualsiasi silenzio e da qualsiasi tentativo di sottrarsi al dovere di chiarire. Pertanto, tramite lei, signor

ho deciso di fare questo intervento poiché questa mattina a Reggio Calabria, di fronte alla sede del Consiglio regionale, si è tenuto un *sit-in* degli operatori socio-assistenziali per lo stato in cui versa il *welfare* calabrese. La legge regionale n. 23 del 2003, in attuazione della legge quadro n. 328 del 2000, nata per risolvere i problemi inerenti al disagio sociale, disturbi del comportamento, disabilità, riadattamento e ad oggi rimane un groviglio inestricabile, a causa dei continui interventi legislativi della Giunta regionale. La conseguenza è stata che tanti destinatari di servizi sociali essenziali oggi subiscono l'immobilismo della Regione Calabria, refrattaria a qualsiasi risposta ai bisogni dei cittadini. Anche oggi la risposta a chi manifestava è stata "picche", eppure i fondi ci sono, ma non arrivano ai Comuni per un contenzioso, oggi finito al Consiglio di Stato, nato per il riparto. Le strutture prive di sovvenzioni rischiano di non poter fornire il vitto alle persone ospitate, per non dire che il personale non riceve lo stipendio da ben dieci mesi. In Calabria non esistono in numero sufficiente strutture che si prendano cura dei soggetti autistici, abbandonati a se stessi se non hanno i mezzi economici per costose trasferte. È il caso di Saverio Corasaniti, diciottenne primogenito di una famiglia catanzarese con grave disagio economico, costituita da padre, madre e altri quattro figli. Niente sostegno alla famiglia, niente assistenza per il ragazzo, nessun centro disponibile a riceverlo e a offrirgli un trattamento di riabilitazione e di mantenimento. Il ragazzo, che non frequenta più la scuola, è regredito e la sua condotta, sempre più difficile da gestire, grava unicamente sui suoi genitori. Da mesi cerco di sensibilizzare gli enti locali e le poche strutture esistenti con interminabili liste d'attesa, senza alcun esito. Questo rapido *excursus* serve ad introdurre questo consesso alla drammatica situazione della Calabria, una Regione ricca di potenzialità e di risorse, che una gestione fallimentare della politica, di destra e di sinistra, ha ridotto in stato di estremo bisogno, privando i cittadini del diritto alla salute, all'assistenza e ai servizi sociali.

poiché i soldi che arrivano o non si sanno gestire o si usano per cattedrali nel deserto, per favorire amici e compari, o si impiegano ad orologeria, in vista delle tornate elettorali, per rinnovare i rapporti di clientela con nuovi contratti di precariato, ma mai per offrire servizi efficienti ai cittadini e opportunità di sviluppo.